nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, l'appuntamento del Consiglio europeo rischia di riprodurre un rituale e una liturgia fin troppo visti negli ultimi mesi. Si tratta del terzo appuntamento del Consiglio europeo in un mese, con un ordine del giorno che è sostanzialmente lo stesso. Indice, dunque, di un problema di malfunzionamento di metodo, prima ancora che di merito, che l'Italia non ha mancato di far notare nel corso delle ultime riunioni, sia nelle sedi istituzionali, cui partecipano i rappresentanti del Governo, che in sede tecnica, a cui partecipano gli *sherpa*. Il metodo, infatti, in questo caso è sostanza. Se il Consiglio europeo si riunisce quattro volte l'anno e assume decisioni che vengono poi implementate e attuate nel corso delle settimane è una storia. Se, viceversa, il Consiglio europeo si riunisce ogni venti giorni producendo documenti sulla cui redazione si perdono le giornate, ma sulla cui implementazione poi si segna un risultato prossimo allo zero il problema del funzionamento va posto non da parte degli euroscettici ma da coloro che vogliono bene alle istituzioni europee e pongono questo tema come cruciale. Apro su questo una parentesi che, però, affronta di striscio la questione della composizione del Consiglio europeo. Un grande studioso ha scritto, qualche mese fa ormai, un pregevole articoletto sulla vetocrazia. Credo che ora stia completando un libro. È uno È uno studioso americano che già ha avuto modo di essere molto analizzato nel corso degli ultimi anni. L'idea del potere di veto, cui non corrisponde un potere decisionale, non riguarda soltanto le istituzioni europee ma anche alcuni Governi europei. Cerco di essere molto breve ed esplicito. Quando abbiamo iniziato a discutere in questa Assemblea la legge elettorale - allora avevamo idee diverse e probabilmente anche adesso continuiamo ad averle -

Stiamo vedendo in queste settimane che la Spagna rischia di non essere in condizioni di produrre un Governo, tanto che non è più esclusa l'ipotesi di un ritorno al voto. In Irlanda e in Slovacchia la situazione elettorale delle ultime settimane non ha prodotto un Governo chiaro e, se volete, in Portogallo il partito uscito vincente dalle elezioni non è quello a cui è stato affidato il compito di formare un Governo. Se a ciò si aggiunge che la Grecia ha votato tre volte in un anno nel 2015 (due volte per le elezioni politiche e una volta per un *referendum*), ci rendiamo conto che il quadro delle regole del gioco e del metodo di lavoro non è uno strumento di discussione per addetti ai lavori ma in Europa è parte del problema che stiamo affrontando. È una grande questione di metodo. Io credo, come ha scritto qualcuno oggi su un importante quotidiano italiano, che alla luce di questo anche chi critica l'Italicum debba riconoscere che l'Italia si accinge ad avere una visione molto più stabile e chiara, come peraltro hanno i francesi e quelli che fanno riferimento a un ballottaggio che, alla fine, per forza dichiara un vincitore. a fronte di un voto non corrisponde un impegno da parte del Governo o comunque del potere esecutivo, il rischio è riprodurre, in misura sempre maggiore, un sentimento di disconnessione tra i cittadini e le istituzioni che produce, come prima conseguenza immediata, l'allargamento della frattura tra cittadini e classe dirigente. questo perché la discussione sul modello di realizzazione e gestione dei Consigli europei non riguarda, come banalmente è stato riportato, anche forse per un eccesso di sintesi da parte nostra, il non voler fare un Consiglio europeo ogni quindici giorni - che pure ha un suo perché ma l'idea stessa di un meccanismo che rischia di impantanarsi sul potere di veto. Si passano i pomeriggi a discutere le virgole, ma alla fine la conclusione è che le decisioni prese non si implementano. Fa da contraltare a questo ragionamento l'ordine del giorno del Consiglio europeo: lo stesso delle ultime volte. E, quindi, anche questo mio intervento non potrà che ripetere i punti fondamentali e qualificanti l'azione del Governo italiano, *in primis* sulla grande questione migratoria. Per utilizzare una sintesi estrema, l'Italia è favorevole all'accordo con la Turchia, ma non a tutti i costi. Ci sono dei presupposti politici, morali e di valore che richiamano la necessità di non venir meno all'ideale costitutivo l'identità europea. Se vogliamo essere sinceri con noi stessi - ci è già capitato in quest'Assemblea in un recente dibattito - l'Italia è un Paese che si può permettere la virtù della coerenza nei rapporti con la Turchia,

sostanzialmente identica (possiamo anche togliere l'avverbio sostanzialmente): apertura vera. Ciò avveniva - ricordo una visita dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad Ankara nel 2009 - in un quadro in cui si cercava di valorizzare lo sforzo che la Turchia stava facendo. L'Italia non ha cambiato posizione, mentre gli altri Paesi europei sì, prima imponendo uno *stop* frettoloso a quel processo di allargamento, a quel dialogo e a quel compiuto negoziato e, poi, insistendo per cambiare immediatamente posizione.

valorizzassimo un gesto molto importante, compiuto qualche ora fa dal nostro Presidente della Repubblica che, nel corso della visita di Stato che sta svolgendo in Africa, tra Etiopia e Camerun, ha scelto di visitare in Etiopia un campo profughi composto non da qualche migliaia di persone, ma da decine di migliaia di persone. Ciò è il segno evidente che l'emergenza migrazione può essere attenzionata dai *media* soltanto in alcune zone del mondo, di una grande emergenza che non tocca soltanto la Turchia, la Giordania o il Libano, ma va dall'Africa al Sud-Est asiatico. Dunque, la posizione dell'Italia sulla migrazione è la stessa della volta scorsa, cioè una posizione coerente. Due anni fa ci dicevano che soltanto noi dovevamo affrontare la questione della migrazione, mentre oggi la realtà dei fatti dimostra che c'è bisogno di una risposta europea. Quando un anno fa, ad aprile, dopo i tragici fatti del Mediterraneo, siamo andati a chiedere una riunione straordinaria del Consiglio europeo, ci hanno guardato come quelli che chiedevano chissà che cosa, ma alla fine la conclusione è che la nostra posizione di allora (cioè che la migrazione è un grande tema europeo e l'Europa deve rispondere) è diventata oggi patrimonio condiviso da tutti. Tuttavia, la risposta ancora stenta ad assumere i contorni di una risposta credibile. Si sono fatti gli *hotspot*, ma non si sono fatti i rimpatri né le *relocation*. Si sono fatti passi in avanti di natura politica, ma allo stesso tempo non si è preso atto che il muro della paura, che è stato costruito, è sempre più forte e che sarebbe sbagliato definirlo semplicemente e banalmente populismo o demagogia, perché si tratta di un sentimento, un seme che sta attraversando tutta Europa e, se guardiamo le elezioni primarie in America, non si ferma in Europa: è il votare sulla base della paura dell'altro, del diverso; è il votare sulla base del terrore di ciò che l'altro può esprimere. Ho parlato dell'immigrazione, della posizione italiana; mi sia consentita una brevissima chiosa, prima di passare al tema economico, su un fatto. Negli ultimi giorni non c'è stata soltanto la vicenda turca, ma gli attentati e la minaccia terroristica hanno colpito al cuore alcuni Paesi, in particolar modo dell'Africa. Faccio riferimento soprattutto alla Costa d'Avorio, dove un *resort* è stato colpito, con i suoi ospiti che sono diventati vittime. Faccio riferimento alla scia di sangue che collega ormai costantemente e settimanalmente zone diverse del nostro pianeta, pianeta, unite dal disegno criminale e atroce di chi vuole disintegrare la nostra vita e, quando non ce la fa, vuole costringerci alla paura. È la minaccia del terrorismo estremista di matrice islamica, che trova le sue vittime e i suoi *target* in un hotel di lusso, in un ristorante a Parigi, in una scuola in Pakistan, in un'università in Kenia, in un museo in Tunisia, in una chiesa in Nigeria. E voglio sottolineare quella bellissima lettera delle quattro suore cattoliche uccise nello Yemen, nel silenzio generalizzato, che fa riflettere chi ha avuto modo di leggerla Sono le sinagoghe, che vengono prese di mira a Bruxelles come a Copenaghen. Il terrorismo non ha finito di compiere il suo disegno terribile, tragico e atroce. Noi dobbiamo convivere con questa minaccia.

noi abbiamo sempre convissuto con l'emergenza e che non è vero che l'emergenza arriva oggi. Ho quarantuno anni. Quando andavo al liceo, la mafia metteva le bombe nelle nostre città. Ricordo perfettamente, un mese prima della maturità, lo scossone, nella mia Firenze, legato a quella Fiat Fiorino e all'attentato agli Uffizi, ai Georgofili, con la morte dello studente spezzino e della famiglia Nencioni. Ma, allo stesso modo, tutti noi abbiamo ben presente dove eravamo quando Giovanni Falcone o Paolo Borsellino venivano uccisi, qualche mese prima; sono quei momenti in cui ti ricordi perfettamente cosa è accaduto e dove eri. Quando si dice: «Me lo ricordo bene, perché quando è arrivata la notizia ero lì», è il segno che quell'evento della storia ci ha tatuato qualcosa nell'anima. La mia generazione dunque è cresciuta con questa minaccia. La generazione di mio padre all'università vedeva i magistrati, i professori e gli studenti spararsi per le strade:

Lasciatemelo dire oggi, 16 marzo, trentotto anni dopo quella terribile strage di via Fani in cui il presidente Aldo Moro fu rapito e gli uomini della sua scorta furono barbaramente trucidati. L'Italia di allora L'Italia di allora viveva una pagina terribile.

era la guerra in Francia, era la guerra in Grecia, altro che Consiglio europeo, altro che discussione sulle virgole. Insomma, la minaccia ha sempre accompagnato la storia del nostro Paese. Oggi la minaccia è diversa. È diversa nelle forme con le quali si manifesta. Penso segnatamente alla scelta di obiettivi e di *target* terribili. Penso anche - lo dico da cittadino europeo

Quella mamma, cittadina europea, nelle periferie di Bruxelles, ad un chilometro e mezzo da dove ci riuniamo per approvare i nostri documenti nei Consigli europei, non soltanto non si era resa conto di ciò che stava avvenendo, ma nell'intervista ha detto una cosa che, personalmente, mi ha molto colpito, ovvero che, se avesse capito cosa stava succedendo, se fosse stata aiutata e se avesse avuto delle istituzioni o dei luoghi del volontariato in grado di aiutarla a cogliere e a scorgere i segni, suo figlio non avrebbe fatto quella fine. Tre mesi dopo la partenza, una telefonata annunciava infatti ai genitori che quel ragazzo, che aveva cambiato nome, era morto da martire. Un cittadino europeo, come cittadini europei sono coloro che hanno fatto

la riduce ad un tema da "spararsi addosso" nei *talk show*, la strumentalizza senza avere la forza di una risposta organica, commette l'errore più grave che può fare un politico: un errore di superficialità e di demagogia. su questi punti, tutte le forze politiche possano accettare il principio che l'Italia ha espresso: un euro in sicurezza e un euro in cultura,

Ho ragione di credere che vi sia lo spazio per portare ad una condivisione anche gli amici dell'ALDE e del PPE. Penso che, se ciò avvenisse, sarebbe finalmente un tentativo di presentare la risposta europea, non soltanto come una risposta securitaria, ma innanzitutto come una risposta culturale. Esiste infine un ultimo punto di discussione, quello legato alla crescita. Ci avviciniamo al prossimo Consiglio europeo con l'ennesimo importante intervento della Banca centrale europea. La Banca centrale europea e il suo Presidente stanno esprimendo una posizione molto seria

che la pericolosa minaccia della deflazione, ormai di casa e residente in Italia e in Europa, non può essere sconfitta soltanto con la via monetaria. Occorre avere la forza di sostenere necessità di una diversa politica di investimenti e di infrastrutture e di restituire denaro e potere d'acquisto abbassando la pressione fiscale. Se si vuole recuperare la sfida contro la deflazione, non si può fare altro che tornare agli investimenti, pubblici e privati, e ridurre la pressione fiscale, in particolar modo delle famiglie e dei consumatori. Come sapete, questi sono i due principi che animano la politica economica del nostro Governo, anche con alcune discussioni in Abbiamo una grande questione relativa a investimenti e infrastrutture. Negli ultimi anni l'Italia ha perso delle posizioni: fino al 2006-2007 l'Italia investiva fino a 40 miliardi di euro sulle infrastrutture pubbliche. Si può discutere di quanto questi investimenti fossero corretti o meno, di quanta necessità vi fosse di interventi diversi, ma il dato di fatto era che l'Italia investiva fino a 40 miliardi di euro,

tagli sulla strada da rimettere a posto di lì a tre anni che non sui servizi, perché tagliare i servizi crea un problema di consenso.

È del tutto naturale e fisiologico che questo si sia poi verificato in virtù anche di alcune strozzature nel sistema della pubblica amministrazione italiana: penso al dissesto idrogeologico, alle bonifiche, alle opere incompiute. Se si hanno miliardi di euro fermi perché non si riesce a far partire dei lavori in quanto per ogni bando di gara ci sono tre ricorsi, è del tutto logico e fisiologico che quei soldi, in teoria appostati, non vengano spesi. Pertanto, la doppia operazione sbloccare gli investimenti e la parte infrastrutturale per i Comuni (questa è stata l'operazione del 2016 con la sostanziale fine del patto di stabilità)

anche per i miliardi di euro bloccati in Sicilia nelle strade, ma anche per il dissesto idrogeologico o per le bonifiche, in alcuni casi anche Questo lavoro italiano, che è un'assoluta priorità, è però quello che serve anche all'Europa, la quale oggi vive con sofferenza la mancanza di investimenti pubblici e privati che il piano Juncker sta cercando faticosamente di sbloccare, ma che sarebbe sicuramente agevolata dal rispetto delle regole che anche altri Paesi dovrebbero mantenere e porsi come obiettivo. Se, ad esempio, i nostri amici tedeschi portassero il proprio *surplus* commerciale dal 7,6 per cento al limite previsto dalla vigente normativa europea del 6 noi avremmo circa 38-40 miliardi di investimenti pubblici che sicuramente aiuterebbero non soltanto la Germania, ma tutta l'Europa. Ecco perché questo primo elemento sulla crescita è legato agli investimenti. Dall'altro lato c'è il tema della flessibilità. Abbiamo già avuto modo di discutere - e vado a terminare - nel corso del nostro dibattito e della replica, le considerazioni legate al *fiscal compact*, al Patto di stabilità e alla flessibilità ad esso connessa. Io trovo che sia importante che l'Italia rispetti la traiettoria. Sono molto fiero e orgoglioso che questo sia l'anno in cui l'Italia non soltanto raggiunge il migliore risultato in termini di *deficit* degli ultimi dieci anni - il migliore ma anche che la curva del debito, stabilizzata rispetto al PIL nel 2015, possa finalmente tornare a scendere a partire dal 2016, perché questo è giusto. L'intensità di tale traiettoria è considerata una variabile della flessibilità. Se si aderisce al *fiscal compact* e lo si segue così com'è, senza flessibilità, la curva è molto ripida, ma la mancanza di flessibilità ti porta ad operare interventi che non sono chirurgici, ma sono interventi di macelleria. Se, viceversa, afferma la flessibilità come valore, e quindi si abbassa la traiettoria senza cambiarne la direzione, è del tutto evidente che ci si può permettere di fare una cosa, probabilmente l'unica che serve in Italia e in Europa, cioè abbassare le tasse, in particolar modo ai consumatori. Gli ottanta euro, l'IRAP sul costo del lavoro, l'operazione che abbiamo fatto sull'IMU e TASI sulla prima casa, ma anche sull'IMU agricola e l'IRAP agricola, non sono operazioni *spot* a fini elettorali, per di più in un contesto in cui, sveliamo questo segreto, non si va ad elezioni. Questo bisognerebbe anche spiegarlo: ci sono gli *spot* elettorali quando ci sono le elezioni e le prossime elezioni, compatibilmente con il rispetto della vigente normativa (e quindi deciderà il Presidente della Repubblica), saranno nel febbraio 2018. Da qui al 2018 sai quante se ne sono scordate di tasse ridotte i cittadini?

la scelta di un certo modello economico e la gestione di una politica di rigore e di *austerity*, è del tutto evidente che le famiglie non reggono. E se è vero, com'è vero, che in Italia gli ottanta euro, l'IRAP sul costo del lavoro, l'IMU e la TASI sulla prima casa, l'IMU agricola e l'IRAP agricola sono delle realtà,

Sono ancora pochi rispetto a quelli che servono, ma sono anche molti di più di quelli che erano attesi. Tutto questo mi porta a dire che c'è una direzione di politica economica indicata da questo Governo che può essere apprezzata o meno ma che, a mio avviso, è la direzione di politica economica di cui ha bisogno l'Italia, di cui ha bisogno l'Europa: ridurre le tasse e fare gli investimenti. Per ridurre le tasse occorre la flessibilità perché senza la flessibilità, dopo aver fatto 25 miliardi di *spendig review* le tasse non le riduce nemmeno mago Merlino. Senza la flessibilità la riduzione delle tasse sarebbe impossibile. Vi è, poi, una grande operazione sulle infrastrutture. Jean-Claude Juncker è stato eletto su questa base: flessibilità e infrastrutture. Un accordo che ha visto insieme il PPE, l'ALDE e il PSE. Il fatto che nel vertice di Parigi il PSE abbia scelto questa come la strategia non dell'Italia, ma del Partito socialista europeo ci rende, a mio giudizio, più forti nella battaglia che dovremo affrontare nelle prossime settimane, perché se qualcuno pensa che basterà la manovra bazooka mensile del presidente della BCE per sconfiggere la deflazione, deve sapere che la BCE sta facendo un grande lavoro, ma senza la politica non si riparte; la BCE fa un grande lavoro ma senza le istituzioni politiche europee l'Unione è finita. E allora, dal nostro punto di vista, andiamo al Consiglio europeo, l'ennesimo, con la forza dei risultati raggiunti (i 16 miliardi di flessibilità conquistata, l'agenda migratoria cambiata), ma al tempo stesso con la consapevolezza che quando questi temi diverranno patrimonio condiviso dell'Europa, solo allora, finalmente, potremo ricominciare a correre.

Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del Presidente del Consiglio e mi sembra strano perché negli scorsi interventi svolti sempre in vista del Consiglio europeo Renzi ci aveva illustrato un mondo che effettivamente a questo punto non c'era. Durante il semestre europeo renziano sembrava si fosse risolto il problema dell'immigrazione e che finalmente vi fossero questi 315 miliardi di investimenti che sarebbero subito giunti dal piano Juncker suggeriti proprio

per suggerire al*Premier* di liberarsi magari di questi gufi che vede intorno - che poi invece bisognerebbe lasciare al loro posto - e dirgli che quando parla di gufi parla di persone che porterebbero sfortuna al nostro Paese

Mi piacerebbe anche parlare del *deficit* al 2,7 per cento quest'anno: bene, era programmato nei suoi documenti, che devono avere una logica. Nel DEF 2014, che ha siglato lei, era programmato al 2

Purtroppo, addirittura l'Europa parla di un'Italia renziana che frena l'economia dell'intera Europa. Di questo dovremmo parlare: delle cose reali, perché lei plaude anche all'operazione di Draghi, però sarebbe interessante anche dire che (a parte il fatto che non è l'ultima, e che le operazioni di Draghi

siamo. Quello che si dovrebbe portare finalmente è un nuovo strumento in Europa, un nuovo strumento che consenta veramente di far arrivare questi 80 miliardi, perché è impossibile pensare che al mese si stampino 80 miliardi di euro e che non arrivino poi agli investimenti

dalla decontribuzione all'IRAP, ai fondi di coesione e sviluppo, dai quali sono stati scippati 3,5 miliardi dei 12, che sono serviti alle grandi imprese per fare solo mere trasformazioni. Per il bene del nostro Paese il Movimento 5 Stelle c'è ed è ben presente: porti questo nuovo strumento,

quando in realtà, purtroppo, lei stesso, con la sua azione - perché è lei che governa - la sta riducendo a fanalino di coda dell'Europa. Il nostro Paese merita molto di più; merita un'azione di governo meritevole quanto lo sono tutti i cittadini. Basta pensare alle banche, basta pensare al padre della Boschi, basta pensare agli amministratori basta pensare agli amministratori che hanno truffato i poveri cittadini! Pensi alle famiglie e alle imprese, agli operai ed agli impiegati: loro hanno bisogno dell'aiuto!

è prevista la celebrazione dei sessant'anni del Trattato di Roma, che fece sognare molti: ebbene, rischiamo di celebrare un drammatico fallimento.

a che l'Europa realizzi una vera politica dell'immigrazione, noi, i nostri figli ed i nostri nipoti avremo molti e seri problemi.

È indispensabile che l'Europa trovi compromessi alti, ma realistici e veri e non si limiti ad approvare documenti

Penso che l'Europa debba andare avanti: siamo in mezzo al guado e se non si va avanti e non si realizza una Europa realmente unita prevarranno, come stanno prevalendo in questo momento, spinte demagogiche che faranno male a tutti noi.

penso che la nostra forza e la nostra credibilità sarebbero maggiori se il Governo riuscisse a fare quello che è difficilissimo da realizzare (e su cui su cui mi sembra si sia fatto ancora troppo poco). Mi riferisco cioè al contenimento della spesa pubblica, al contenimento degli sprechi, alla riduzione degli enti inutili, che sono ancora tanti, troppi e che non si riescono a ridurre. capisco non sia facile, però troppi soldi del contribuente italiano sono sprecati e si disperdono in mille rivoli

Credo che se noi riuscissimo a realizzare qualcosa, non solo porremmo le premesse per ridurre le tasse, non a debito, ma mettendo a posto i conti, ma anche la nostra credibilità nel fare la voce grossa e nel portare avanti le nostre istanze sarebbe maggiore. Questo penso su questo argomento. Ripeto: io sono vecchio, sono nato quando cominciava la guerra, ho festeggiato nel 1957 il Trattato di Roma, ho viaggiato con il passaporto, poi con la carta d'identità e ora viaggio liberamente. Io non mi rassegno e nessuno di noi si deve rassegnare al fatto che si torni indietro, perché sarebbe troppo triste per noi, ma soprattutto grave

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio, troppe volte l'Europa ha ignorato le immagini che arrivano dai suoi confini; sono immagini di un'umanità in cammino, che cerca riparo da guerre e terrorismo, che sono i nostri stessi nemici. Sono intere famiglie, tantissimi anziani, donne, bambini, che lasciano città distrutte, vite spezzate di intere generazioni di siriani, di afghani, di libici, tanti giovani che provengono dai Paesi del Corno d'Africa, del Sub-Sahara. Quella stessa avversità è toccata a molti europei, che settant'anni fa hanno cercato riparo altrove, altrove, costretti a lasciare le case in macerie, sventrate dalla guerra e dalla fame. I più massicci flussi migratori della storia dell'umanità sono stati compiuti dagli europei. E se noi perdessimo la memoria di tutto questo, se perdessimo il vissuto delle migrazioni, del ricongiungimento tra europei dell'Est e dell'Ovest, del Sud e del Nord, perderemmo, signor Presidente, la nostra stessa identità, il collante e i valori che ci tengono insieme. Eppure questo è quello che sta accadendo. Le sfide globali si ingigantiscono l'Europa, invece, tende a rimpicciolirsi, a rinchiudersi, rincorrendo egoismi, opportunismi; è quella globalizzazione dell'indifferenza senza responsabilità sociale, di cui Papa Francesco, in maniera quasi profetica, parlò a Lampedusa, qualche mese prima della tragedia del 3 ottobre 2013. Ci sono in Europa disuguaglianze insopportabili, che hanno svuotato le nostre democrazie; politiche economiche sbagliate, perché ormai è chiaro che l'austerità e l'europeismo sono nemici. Per questo hanno avuto e hanno buon gioco i populisti e i nazionalisti ad ingigantire la paura della crisi con la paura delle guerre, delle migrazioni, del terrorismo: i Le Pen, gli Orbán, i Farage, i Salvini, i Grillo *(Commenti dal Gruppo M5S)*, che fanno riemergere quel demone del nazionalismo che noi pensavamo sconfitto negli anni Trenta, che tanta distruzione ha portato nel nostro Continente. Muri e filo spinato saranno la fine la fine dell'Europa e senza Europa i più deboli saranno ancora più deboli, i più forti ancora più forti. Il fenomeno migratorio che abbiamo di fronte è sideralmente diverso da quello che abbiamo vissuto negli anni Ottanta e negli anni Novanta. Quello attuale è un fenomeno che segna la nostra epoca, è uno spartiacque epocale e ha innanzitutto una natura politica. Basti pensare a quello che è successo solo pochi anni fa, nel 2011: le grandi speranze accese dalle cosiddette primavere arabe, che nel volgere di soli pochi mesi si sono trasformate nel dramma dei barconi che attraversavano il Mediterraneo, gestiti dai trafficanti di schiavi, a loro volta assoldati dai capataz delle grandi organizzazioni criminali internazionali. questa immigrazione nasce innanzitutto dalla frantumazione dell'ordine politico tra l'Africa mediterranea e il Medio Oriente con i suoi focolai più virulenti nelle guerre civili in Libia, in Afghanistan, in Siria, in Yemen. L'Europa non può far finta di nulla, anche perché l'Europa e l'Occidente hanno precise responsabilità su quello che è successo. Oggi tocca ad una nuova classe dirigente riscattare errori, tocca ad una nuova generazione di europei fare fino in fondo la propria parte. L'Europa troppo a lungo ha fatto finta di non vedere, concentrando tutte le sue energie verso il partenariato orientale come se fosse possibile per l'Europa per l'Europa fare a meno del Mediterraneo: non è possibile un'Europa senza Mediterraneo. qui in quest'Aula abbiamo fatto diventare ricorrenza e memoria nazionale, l'Europa balbettava, nonostante campeggiassero su quella spianata di Lampedusa centinaia di bare e alcune di esse fossero bianche perché erano bare di bambini. È toccato all'Italia allora fare un passo decisivo, riscattare la dignità perduta di un intero continente europeo; riscattare anche l'ignominia di una legge, la cosiddetta Ed è merito anche di due anni di iniziativa politica di questo Governo, a partire dal semestre europeo a guida italiana, se l'Europa oggi comincia ad avere, anche se è ancora fragile e incompleto, un primo nucleo di politica comune sull'immigrazione. Senza una politica dell'immigrazione non è possibile avere una comune politica estera: le due cose sono inscindibili e fondamentali entrambe. L'Europa faccia l'Europa con politiche di accoglienza, di integrazione, di sicurezza, che le daranno quella legittimazione morale che è imprescindibile per poter avere la piena legittimazione della politica, per imporre soluzione ai conflitti in Medio Oriente. Va recuperato molto terreno perduto come quello del dialogo con la Turchia che lei richiamava. Oggi la Turchia è un *partner* indispensabile per gestire la vicenda migratoria, ma ribadendo, come lei ha detto, alcune condizioni inderogabili sulle quali ci richiamano importanti organizzazioni non governative: il rispetto dei diritti umani, il rispetto del pluralismo e della libertà il rispetto delle prerogative della minoranza curda. E se abbiamo costruito successi militari contro l'ISIS, dobbiamo ringraziare anche quello sforzo enorme che questa minoranza sta facendo. È una situazione complicata anche dal dal fallimento ormai conclamato delle regole che abbiamo sull'asilo. Serve un diritto di asilo europeo, serve archiviare quel Regolamento di Dublino che impedisce ai rifugiati che arrivano di lasciare il posto di prima accoglienza per raggiungere le proprie destinazioni. E noi abbiamo cominciato a farlo con la regola del ricollocamento nei Consigli europei della primavera di un anno fa, che sono seguiti anch'essi a una tragedia enorme, quella dell'aprile 2015, al largo del canale di Sicilia, con quasi 900 morti. Quella ripartizione significa nei fatti archiviare Dublino; quella ripartizione deve esserci subito perché ancora concretamente non la si vede. È necessario tagliare i fondi a quei Paesi che non prendono i rifugiati contravvenendo alla regola costitutiva dell'Europa: essere solidale oppure non essere. Questo permetterà anche la politica dei rimpatri, perché Schengen Dublino sono in contraddizione. Allora è giusto che per salvare Schengen sia definitivamente archiviato il Regolamento di Dublino. Vanno poi aiutate le economie africane nel Mediterraneo. Basta un attentato che porta con sé non solo dolore, ma morte e sangue,

per la ripresa economica. Questo è fondamentale. Se ripartono quelle economie, sarà un modo per arginare i flussi verso l'Europa. E poi, signor Presidente, voglio dire che c'è un esempio italiano importante, un primo esempio italiano che può essere di scuola per l'intera Europa. Il 29 febbraio sono arrivati in Italia, a Fiumicino, 93 siriani, grazie all'accordo tra alcune ONG, quali la comunità di sant'Egidio e la chiesa valdese. Con il supporto del Governo italiano si è aperto per la prima volta un corridoio umanitario che consente di mettere in salvo salvo chi scappa dalla guerra rispetto ai trafficanti di schiavi e di morti, di mettere gli Stati dalla parte di chi bussa e non di chi chiude le porte, di salvare chi fugge dalla guerra e di aiutare chi ha diritto e, invece, di rimpatriare chi quel diritto non lo ha. Questo esempio di corridoio umanitario, di ponte da costruire, sia esempio per tutta l'Europa. i morti a largo di Lampedusa o di Bodrum sono morti europei. Così come i ragazzi in fondo al Mediterraneo sono gli stessi ragazzi rimasti uccisi al Bataclan o davanti alla fermata del bus di Ankara. Per questo è importante costruire sicurezza con l'integrazione. Per questo è importante puntare sulla cultura, sul risanamento delle periferie come luogo principale di prevenzione. Per questo sta a noi costruire una nuova classe dirigente europea che combatta la diseguaglianza, che riesca, in questa temperie, a tener tener viva la spinta di una società aperta e inclusiva. Signor Presidente, due immagini in particolare ci hanno colpito, soprattutto se le affianchiamo. Una è l'immagine di Aylan, il bambino l'altra è l'immagine del bambino, pieno di vita, tra il fango della tendopoli di Idomeni, tra Grecia e Macedonia.

affinché davvero si compia uno sforzo per fare in modo che la vita vinca sempre sul fango. che il Presidente del Consiglio si lamenti del malfunzionamento del Consiglio europeo a noi, sinceramente, interessa poco. A noi interessava sapere quali posizioni vorrà assumere il Governo italiano rispetto alle gravi crisi chiamato ad affrontare. Il presidente Renzi, come suo solito, non ha detto assolutamente niente. Il vuoto totale. Il nulla assoluto. È davvero triste che abbia fatto ricorso all'espediente di citare le vittime di via Fani e Falcone e Borsellino

17 e 18 marzo si discuterà principalmente di ulteriori misure per affrontare la crisi migratoria e dei rifugiati. Si discuterà, in particolare, delle richieste avanzate dalla Turchia per collaborare con l'Unione europea nella gestione di tali flussi. Cosa chiede la Turchia all'Unione europea per collaborare? Tre miliardi di euro in più, dopo quelli recentemente concessi; la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi in viaggio verso l'area Schengen europea; l'accelerazione della procedura di ingresso della Turchia nell'Unione europea. Queste sono le tre richieste e su questi tre punti non abbiamo sentito nulla da parte del Presidente del Consiglio. Nella nostra risoluzione, molto modestamente, abbiamo svolto alcune considerazioni rispetto a queste istanze. La prima è che chiedere altri tre miliardi, dopo averne appena ottenuti altrettanti, rappresenta una evidente manifestazione di inaffidabilità da parte del Governo turco, sta giocando al rialzo senza nessuna garanzia che intenda realmente collaborare con l'Unione europea per limitare i flussi migratori provenienti dalla Siria e dai Paesi limitrofi. Allo stato attuale, la Turchia si è intascata i soldi dei cittadini europei, ma non ha migliorato in alcun modo il controllo delle frontiere. In questi primi mesi del 2016 sono giunti in Grecia dalla Turchia ben 126.000 migranti. è che la liberalizzazione dei visti dalla Turchia potrebbe rappresentare un ulteriore rischio di ingresso di terroristi in Europa e in Italia e va quindi scongiurata. In questa fase storica non è semplicemente prematuro. Rappresenterebbe una gravissima imprudenza e un atto irresponsabile. Vengo al terzo punto. La richiesta di accelerare l'ingresso della Turchia nell'Unione europea è semplicemente irricevibile. Per la Lega Nord lo è a priori, ma oggi, nelle condizioni attuali, lo dovrebbe essere per tutti.

Il flusso attraverso il proprio territorio di uomini e donne che intendono arruolarsi nel sedicente Stato islamico non è controllato, anzi sembra tollerato dalle autorità turche. La Turchia attacca militarmente i curdi che rappresentano gli oppositori più impegnati nella lotta contro l'ISIS. Vorremmo ricordare che, se anche Cipro è un piccolo Stato dell'Unione europea, il rispetto nei suoi confronti va tutelato dagli altri Paesi, compresa l'Italia. In queste ore le autorità turche hanno confermato la loro indisponibilità a riconoscere Cipro come stato indipendente e sovrano. Allora, Presidente, di cosa stiamo parlando? Il Governo turco è assolutamente inaffidabile. *(Applausi è che il Governo turco manipola i flussi migratori per ottenere contropartite dall'Unione europea sia economiche che politiche. Il presidente Renzi si dia una svegliata. La realtà dei fatti è sotto gli occhi di tutti. Ci permettiamo una raccomandazione: non regali altri soldi dei cittadini italiani alla Turchia. Ha già fatto questo errore. Non si permetta di ripeterlo e la smetta, per favore, con il teatro che continua ad andare a fare in Europa. Racconta continuamente agli italiani che va in Europa a sbattere i pugni sul tavolo, ma allora ci spieghi perché torna in Italia sempre a mani vuote. Torna a mani vuote perché in Europa ha perso ogni credibilità, perché non le dà più retta nessuno. Vediamo ora come si sta comportando il Governo italiano e non l'Europa. Se la politica dell'Unione europea nei confronti delle migrazioni di massa dall'Asia è inefficacie e inconcludente, quella dell'Italia è semplicemente un disastro. L'Europa da mesi si sta occupando esclusivamente del tentativo di arginare il flusso di migranti della rotta balcanica. Dell'arrivo di centinaia di migliaia di clandestini dalla Libia non si occupa più, sempre che se ne sia mai occupata. Ormai è assodato che quello è e rimarrà un problema tutto italiano, aggravato dall'avanzata dell'ISIS. Lei, presidente Renzi, ha speso 3,3 milioni di euro degli italiani nel solo 2015 per ospitare decine di migliaia di giovani uomini stranieri negli alberghi di tutta Italia. presidente Renzi, insieme al suo compagno di viaggio Alfano, ha dato ordine alle prefetture di trovare altri 50.000 alloggi nel corso di quest'anno e qualche suo solerte prefetto è arrivato a minacciare i cittadini italiani di requisire le loro abitazioni perché autorizzato dal Governo. Ma fin dove volete spingere la vostra follia e la vostra arroganza? Presidente, le faccio osservare che in Europa stanno tutti bloccando le frontiere. L'Italia rischia di rimanere l'ultima e unica destinazione per tutti i migranti di Africa e Asia perché dalla Grecia si potranno dirigere solo verso l'Albania e da lì, via mare, in Italia. Lo faranno perché sanno che in Italia c'è un Governo di sprovveduti e sconsiderati. Le vostre parole d'ordine sono semplici: porte aperte a tutti. Presidente, non siamo solo noi dodici senatori della Lega Nord che la pensano così perché ormai, nonostante le sue recenti manovre per occupare la RAI, la maggioranza degli italiani sta aprendo gli occhi. Hanno capito che il suo Governo non sta affrontando l'emergenza migratoria che interessa l'Italia; il suo Governo ne è semplicemente il principale responsabile. I risultati dell'azione del vostro Governo sono sotto gli occhi di tutti: i flussi migratori aumentano e stiamo subendo un'invasione senza sosta. Le domande di asilo, il cui *iter* è peraltro lentissimo, sono quasi tutte rigettate, a dimostrazione che in albergo ospitiamo clandestini e non chi scappa dalla guerra. Siamo gli ultimi in tutta Europa nell'attuare i rimpatri di chi non ha diritto di rimanere in Italia e non controlliamo nemmeno l'identità di chi arriva nel nostro Paese, con buona pace della lotta contro il terrorismo. La politica dell'Italia sull'immigrazione è semplicemente un disastro. Il vostro Governo è un disastro. Svegliatevi dal vostro sogno, perché per gli italiani è un incubo. L'Italia che descrivete in quest'Aula e anche fuori ogni volta che parlate, semplicemente non esiste. È un'illusione. I cittadini vivono nella cruda realtà, che è fatta di paure e insicurezze per il futuro loro e delle proprie famiglie. Si tratta di insicurezze alimentate non, come dite voi, dal nostro presunto e inutile allarmismo, ma dagli atti concreti della vostra azione di Governo. hanno paura di perdere il lavoro o di non riuscire a ottenerlo. L'anno scorso sono emigrati dal nostro Paese 100.000 italiani in cerca di fortuna all'estero. hanno paura nelle loro case perché il Governo non inasprisce le pene per i delinquenti, ma svuota le carceri e penalizza chi osa difendersi. per i mutui sulla casa che fanno fatica a pagare e di un Governo che rende più facile il pignoramento delle abitazioni da parte delle banche affinché possano far cassa. hanno paura di non riuscire ad ottenere una pensione dignitosa per l'infame legge Fornero, votata nel 2012 da quel Partito Democratico di cui lei, signor Presidente del Consiglio - glielo ricordo - è il segretario nazionale. hanno paura che vogliate mettere le mani sulle pensioni di reversibilità e di essere derubati dei risparmi di una vita, che possono sparire dalla sera alla mattina con un decreto del vostro Governo. Questo è il Paese reale in cui stiamo vivendo e non quello delle chiacchiere del parolaio che lo sta guidando. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Un parolaio che non è stato nemmeno eletto dai cittadini e che continua a vendere un ormai insopportabile e stucchevole ottimismo assolutamente ingiustificato e illusorio. concludere. Abbiamo ascoltato per l'ennesima volta il lungo elenco di tutti i suoi successi in Italia, in Europa e nel mondo. Lo abbiamo fatto con la solita pazienza: quella pazienza che gli italiani ormai hanno perso da molto tempo. Signor Presidente del Consiglio, ci permetta un ultimo consiglio disinteressato: torni con i piedi per terra, se le è possibile, e cominci a mettersi in discussione. Tutti noi dovremmo farlo perché fuori da questo Palazzo

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,

utilmente adeguato. In questo senso, mi permetto di sollecitare anche l'attenzione del Presidente della Commissione affari esteri del Senato, l'amico Pier Ferdinando Casini, perché vorrei fornire alcuni elementi di merito

il Ministro dell'interno, l'onorevole Alfano, il 10 marzo scorso ha detto che non esistono evidenze in ordine all'apertura di una nuova rotta adriatica per la migrazione dei richiedenti asilo.

nella Commissione difesa del Senato, il generale comandante della KFOR, l'italiano Guglielmo Luigi Miglietta, ha detto testualmente: «La seconda minaccia è connessa all'enorme flusso di migranti a cui è sottoposta la penisola balcanica. (...) Il rischio si presenta quindi come duplice: i migranti potrebbero entrare da sud (dalla Macedonia), nel caso in cui la Serbia dovesse decidere di chiudere il suo confine meridionale; ma potrebbero anche - e soprattutto - entrare da Est, ossia dai confini serbi, se altri Stati nel Nord della penisola dovessero seguire l'esempio di Ungheria e Croazia, impedendo i transiti. Infatti, i migranti si troverebbero bloccati nei centri di accoglienza in Serbia e ciò potrebbe indurli a tentare la rotta più breve per l'Europa: quella che, attraverso il Kosovo, giunge in Albania e da lì, riaprendo la tratta adriatica, in Italia». del Consiglio, io gradirei che nella sua replica lei ci chiarisse se il Governo è consapevole di questo particolare. È vero quello che dice il Ministro dell'interno, che non c'è alcuna evidenza di una rotta adriatica che porterà i richiedenti asilo dall'Albania in Italia, o è vero quello che dice il comandante di KFOR? Peraltro il comandante di KFOR, cioè il comandante di un contingente NATO, dice di aver ricevuto istruzioni e ordini anche sul piano politico. politico. Dice infatti il comandante Miglietta: «L'azione (...) si è concretizzata nella richiesta ai Paesi partecipanti» - sta parlando dei Paesi NATO - «di un sostegno politico per eventuali azioni di assistenza umanitaria, che non rientrerebbero strettamente tra i compiti assegnati alla forza multinazionale». Miglietta, cioè, dice in audizione che la NATO ha avuto indicazioni per accelerare il percorso dei migranti, mettendo

- e ha ricevuto questi ordini dai livelli politici della NATO. Allora io le chiedo, signor Presidente del Consiglio: andandosi a sedere al tavolo europeo, lei è consapevole di questo? Ed è consapevole che il Governo italiano può aver assentito a questa strategia,

Quali precisi paletti metterà, perché non ci sia il rischio che, nel rimpallo di responsabilità e comunque nell'equivoco su una strategia che debba coinvolgere Unione europea e Turchia, tutto non ricada invece sulle spalle dell'Italia?

del tutto disatteso dagli altri *partner*. E dico questo perché su una cosa lei, signor Presidente del Consiglio, ha pienamente ragione: il vero danno all'Europa non lo fanno gli euroscettici, ma lo fanno quelli che si dicono euroconvinti e si comportano da eurocretini. In questo modo noi destabilizziamo sistematicamente la credibilità dell'Unione europea, e diventiamo soprattutto poco credibili nei confronti dei nostri cittadini. Mi premeva in questa fase del dibattito, prima della dichiarazione di voto, poter porre alla sua attenzione questo passaggio, perché credo che da un giudizio cogente del Governo su questa materia si possa articolare anche la nostra opinione sulle sue comunicazioni. Le ricordo, da questo punto di vista, che nella conclusione che dovrete tirare domani, come Consiglio europeo, sull'accordo con la Turchia non può essere messo da parte cosa avviene della rotta balcanica (intesa come percorso che conduce dalla Grecia fino all'Austria), perché è stata per l'appunto bloccata, per l'appunto bloccata, ma cosa accadrà se ci sarà una leggera deviazione verso sinistra e, se si arriverà in Albania, in Montenegro e da quel momento verso l'Italia, ponendo il nostro Paese ancora una volta nelle condizioni di essere il capro espiatorio di una situazione per molti versi incredibili. *(Applausi

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, ho sentito il Presidente del Consiglio dirci che il Consiglio europeo si riunisce ogni quindici giorni e che i risultati che provengono da quelle riunioni sono pari a zero,

otterremo questi risultati». Poi, grazie al cielo, siccome i numeri non hanno colore politico, se parliamo di migranti, le posso ricordare qualche numero: nel 2012 ci sono stati 13.267 arrivi. Certo, poi le condizioni sono cambiate,

«È un primo passo. Abbiamo completamente coperto il primo anno che riguarda i primi 20.000 ricollocamenti previsti tra Italia e Grecia». E più avanti, si dice ancora. «Tra sei mesi si rifarà il punto della situazione, per vedere se sarà possibile raggiungere comunque l'obiettivo iniziale, che era di 40.000».

Nessuno! Cosa fa, dunque, chi viene qua senza avere un lavoro? O cade vittima del lavoro nero, o entra nel circuito dell'assistenzialismo cronico, che evidentemente è tanto caro al Governo di sinistra, o va a delinquere. intanto le nostre città sono diventate grandi parcheggi della disperazione europea, perché gli arrivi non si fermano, i dati sono in continuo aumento

Lei ci parla di Falcone e Borsellino e mi viene da scattare in piedi quando sento quei nomi, ma oggi i temi sono diversi. Voglio un Paese che guarda avanti e lei deve avere il coraggio di guardare avanti e dirci perché questi numeri non cambiano.

avviene perché costoro vanno in giro per le nostre città, nelle nostre piazze e nelle stazioni, e le persone, quando va bene - uso un eufemismo - vengono disturbate continuamente. Questo Governo non fa nulla e non ottiene neanche quello che avrebbe dovuto essere l'unico grande successo in campo migratorio, che è quello dei ricollocamenti. Quindi, mi aspetto risposte in tal senso, perché i numeri non hanno colore politico. Il tempo a disposizione non mi permette di entrare anche nelle questioni economiche, ma sulla pressione fiscale viene da sorridere, perché i modi della pressione fiscale, signor Presidente, sono diversi. Basta applicare le accise sui vini

Da tempo l'agenda europea comprende sempre gli stessi problemi, sui quali francamente dobbiamo dire che non si sono fatti passi avanti significativi, ma persino dei passi indietro, con uno stallo pericoloso che rischia di peggiorare la situazione. Il punto politico fondamentale è sempre lo stesso: senza un'Europa con una coesa e chiara strategia politica sia in campo migratorio che economico economico si può aprire un vuoto destinato ad essere occupato da quelle forze politiche più estremiste e populiste, sia di destra che di sinistra, come abbiamo visto in Germania qualche giorno fa. l'Europa è posta di fronte a un bivio: o si dimostra capace di promuovere, da un lato, lo sviluppo economico e, dall'altro, di saper governare e gestire la crisi economica, oppure inevitabilmente prevarranno le forze politiche che scommettono sul fallimento della moneta unica e del progetto storico dell'Europa unita. Io credo che l'Italia in Europa abbia le carte in regola più di tutti gli altri Governi, perché fin dall'inizio ha saputo affrontare la questione dei migranti con grande serietà. Lo ha fatto mettendo davanti a tutto il principio fondamentale di salvare le vite, anche quando l'Europa ha girato la testa dall'altra parte, lasciandoci soli ad affrontare un dramma immenso. Sappiamo che, solo quando il problema dei migranti ha investito direttamente l'Europa centrale, esso è entrato davvero a far parte dell'agenda europea con la conseguente richiesta di solidarietà. Eppure, nonostante questo, siamo ancora qui, fermi, con il rischio di uno stallo e persino di compiere irreparabili passi indietro, come potrebbe essere la sospensione del Allo stesso modo, sulle questioni economiche, io credo che l'Italia abbia mostrato una linea coerente e seria. In particolare il suo Governo, signor Presidente, ha cominciato a realizzare riforme importanti, strutturali e necessarie al Paese, ma puntualizzando sempre che la politica di sola austerità non soltanto non funziona, ma rischia di aggravare i problemi della crisi economica.

che si può ottenere solo con il rilancio degli investimenti e la riduzione delle tasse. Dunque, è giusto e necessario consolidare e persino cercare di ottenere maggiore flessibilità, che non significa avere conti sregolati, sregolati, ma avere la giusta autonomia nel fare delle scelte di nuovi investimenti per rimettere in moto il motore dell'economia. Io credo che, se non verrà compreso tutto questo e non diventerà l'obiettivo dell'Europa, perderemo tutti. Non vinceranno nemmeno le forze populiste, perché la loro battaglia è senza futuro. I problemi del mondo, oggi, si possono affrontare solo con un'entità sovranazionale come quella che abbiamo cercato di costruire dal dopoguerra ad oggi. Dunque, non c'è alternativa ad un'Europa unita, ma deve essere un'Europa che funziona, un'Europa che sappia dare risposte concrete. E io credo che l'Italia, signor Presidente, possa essere protagonista di questo cambiamento di rotta, persino di questa rinascita dell'Europa. Concludo, Presidente, dicendo quindi che possiamo e dobbiamo lavorare solo a questa prospettiva, al di fuori della quale c'è solo il ritorno al passato e a politiche destinate a fallire in un contesto globale ormai sempre più difficile e serrato. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, una domanda interessante, che credo meriti una sua risposta in sede di replica, gliel'ha già posta il collega senatore Mauro, a proposito della chiusura di una rotta balcanica che rischia di riaprire l'angoscia di una rotta adriatica che potrebbe riproporsi nelle prossime settimane. però, che sia soprattutto opportuno non perdere di vista la sua considerazione iniziale. Quando da un vertice all'altro, da quattro settimane in là, la soluzione dei problemi è soltanto parziale e si ha la sensazione di una dilazione permanente, appunto al prossimo Consiglio europeo, c'è qualcosa che non funziona istituzionalmente nella costruzione europea. Il collega Carraro, con molta amarezza, ha parlato addirittura di fallimento di un sessantennio di europeismo. Da parte sua, signor Presidente del Consiglio, mi è sembrato invece che l'espressione «vetocrazia», ricavata da una pubblicistica intelligente, sia quella che maggiormente la soddisfa, ma io ho l'impressione che non si tratti di questo. Quella delle migrazioni è un'emergenza delle emergenze. Che senso ha, colleghi del Senato, riempirsi di parole stamattina e farsi tronfi ostentando retorica e moralismo a proposito di alcuni nobili episodi rievocati in un bel film, «Fuocoammare» - lei, Presidente del Consiglio, ne ha fatto oggetto di un omaggio ai colleghi nello scorso Consiglio europeo - e poi cercare di cancellare dalla memoria le immagini degli ultimi telegiornali? L'Europa non è riuscita neanche a edificare una tendopoli appena appena decorosa alla frontiera con la Macedonia. E allora, signor Presidente del Consiglio, accanto a quello postole dal collega Mauro, io vorrei porre un altro quesito: che fine ha fatto quel documento del Ministro degli interni italiano e del Ministro degli interni tedesco cui abbiamo sentito parlare a cavallo con l'ultimo Consiglio europeo? I ministri Alfano e de Maizière si rivolgevano

di tante retoriche di moralismo di massa alle quali capita di abbandonarsi anche in queste Aule. Il documento dei Ministri degli interni si proponeva - a mio giudizio - un percorso possibile e credibile per resuscitare Schengen. Qual è il percorso credibile e possibile per risuscitare Schengen? quello di cui parlavano Alfano e de Maizière: si tratterebbe di trasformare di fatto Frontex in una sorta di polizia di frontiera europea; si tratterebbe di prescindere dal Paese di ingresso nel fissare le quote di redistribuzione tra i singoli Paesi. Questo, collega Verducci, significa andare al di là della contabilità ("Dublino 1, il 2002, l'approvazione; c'era il Governo Letta o c'era già il Governo Renzi", e via dicendo). Se poi riusciamo a risuscitare Schengen in questo modo, fissando delle quote che prescindano dal Paese di ingresso, riusciremo a costruire qualcosa di europeo e di europeista. Sennonché, inevitabilmente, l'iniziativa di Alfano e di de Maizière era diretta al Presidente polacco, a Donald Tusk, e non all'interlocutore vero. L'interlocutore vero è fuori l'Europa ed è la Turchia di Davutoğlu, di Erdogan, se volete; quella Turchia nei cui confronti la politica della Merkel, domani, è in qualche modo obbligata. Si tratterà di chiedere una riammissione di migranti dalla Grecia alla Turchia in cambio del reinsediamento di rifugiati siriani dalla Turchia in Europa. È un modo di limitare il disordine. Verducci, piano, piano con la retorica: benemerita l'accoglienza italiana dei 93 siriani, ma sono 93. Guardate che la Turchia ne ospita - in condizioni tutt'altro che indecenti - 2,5 milioni. Ecco perché quello della Turchia è un problema che inevitabilmente approda nell'agenda europea. Signor Presidente del Consiglio, nessuno più di me è sensibile agli irrinunciabili valori europei, soprattutto inglesi e francesi, della libertà di stampa; la libertà di stampa si lega alla continuità della libertà parlamentare. Quando in Turchia il regime parlamentare muoveva i suoi primi passi; quando la Turchia, forte della lealtà occidentale con la quale era stata nella NATO - si erano fatti chiamare i bulgari della NATO (termine abbastanza sgradevole e sguaiato) bussò all'Europa, l'Europa le disse di no, e glielo disse con tracotanza. Signor Presidente del Consiglio, lei è passato ovattato su quella vicenda, ma in quella vicenda c'è un protagonista, ed è l'allora Presidente della Commissione europea, perché Erdogan non era ancora Presidente del Consiglio, ma soltanto segretario del partito.

mentre proprio quelle amicizie erano la migliore attitudine all'Europa e all'ingresso in Europa della Turchia. la Turchia, sentitasi respinta, ha cambiato completamente politica in una sorta di fuga dall'Occidente, il cui atteggiamento con Israele è la cartina di tornasole. Se noi vogliamo riaprire un discorso con i cosiddetti bulgari della NATO, possiamo farlo soltanto in nome della solidarietà occidentale. E, quindi, non possiamo far vedere che non ci ricordiamo quando, nei giorni della polemica sull'intervento americano in Iraq, il presidente Prodi, con arcigna convinzione, volle chiudere la porta all'ingresso in Europa della Turchia e provocare

sareste stati un grande Paese europeo, come nel sogno di Kemal Atatürk, e vi siete ridotti al rango di piccola potenza di interdizione orientale nel Mediterraneo.

dal presidente egiziano al-Sisi, è a nostro avviso un passo in avanti sulla strada della ricerca della verità sul barbaro omicidio di Giulio Regeni. Siamo, tuttavia, ancora lontani da quel risultato, che sarà raggiunto solo se il Governo italiano sarà inflessibile nel pretendere che i colpevoli di quel delitto siano identificati e puniti ad ogni costo. Anche perché, presidente Renzi, non credo le sarà sfuggito

Non è più differibile - a nostro avviso - una revisione dei trattati europei, a partire dal *fiscal compact.* Bisogna superare l'austerità e non bisogna farlo timidamente

che avvertivamo quando poche voci hanno cercato, in quegli anni, di opporsi a quella sorta di pensiero unico dominante. E, proprio per questo, vorrei continuare a dire con chiarezza

esprimiamo un giudizio molto diverso dal suo, proprio riguardo ai principali provvedimenti del suo Governo, che riteniamo siano stati dannosi o quantomeno inefficaci.

davvero mi verrebbe da parlare di un *flop act* più che di un *jobs act*! Dinanzi a queste questioni fondamentali e urgentissime, penso sarebbe utile fare un bilancio un po' più serio degli anni del suo Governo, ma non lo farò oggi, perché vorrei concentrarmi su un altro tema che la coscienza di ogni persona ci fa sembrare ancora più urgente. Quel terreno - e parlo ovviamente dell'immigrazione è quello su cui davvero si dovrà provare se l'Unione europea è un passo avanti oppure un passo indietro sul piano della civiltà collettiva del nostro continente. Questo fenomeno, che noi molto spesso, troppo sbrigativamente, chiamiamo emergenza e che invece - come ha detto qualche altro senatore questa sera, e ne sono felice è un evento storico di carattere epocale, può essere fronteggiato soltanto a un livello adeguato, e non con le politiche di piccolo cabotaggio e di tamponamento

ad esempio quelle pronunciate dal presidente del Consiglio europeo Tusk, il 7 marzo scorso, dopo la riunione dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea con la Turchia - appaiono - a nostro avviso - non semplicemente inadeguate, ma anche molto inquietanti. Diceva Tusk che Diceva Tusk che tutte le decisioni mandano un messaggio molto chiaro: i giorni dell'immigrazione illegale verso l'Europa sono finiti. Davvero quella frase sembra richiamare un vero e proprio cambio di marcia;

in un approccio che non solo è inumano per i principi (su cui, peraltro, l'Unione si fonda), ma che è anche illusorio, probabilmente addirittura suicida rispetto a quello che accade nel mondo. Gli accordi di Schengen sono stati demoliti nei fatti e lo diventano ogni giorno di più. La stessa frontiera chiusa costringe moltissimi esseri umani ad ammassarsi in condizioni che coprono questo continente di vergogna ogni giorno di più. Non lo so e, quindi, vi chiedo: come può una civiltà considerarsi tale quando assiste impassibile e muta

non colpisce soltanto i migranti, ma si abbatte anche sugli Stati di frontiera, ad esempio sulla Grecia, la stessa che, dopo essere stata strangolata con l'*austerity* dall'Europa, è oggi abbandonata dall'Europa ed è condannata a gestire praticamente da sola una pressione che sarebbe ingestibile per qualsiasi Stato. Naturalmente vale lo stesso anche per l'Italia, che vive una situazione analoga anche se, fortunatamente, almeno nei numeri, meno meno drammatica e meno tragica. Le cifre parlano da sole, le conosciamo bene e ce le siamo dette: dall'inizio dell'anno 141.000 migranti sono sbarcati in Europa; di questi 132.000 hanno raggiunto la Grecia e soltanto 9.000 il nostro Paese. Ma i dati non sono solo questi. L'altro dato drammatico è che le vittime accertate nel Mediterraneo sono già state 444: una strage, signor Presidente, continua e infinita. e infinita. Al cospetto di questa tragedia, la sola via d'uscita che l'Europa civile e democratica è riuscita a immaginare è un accordo con il regime turco;

Nei prossimi due giorni il Consiglio ratificherà un accordo che regala al regime turco altri tre miliardi di euro, il doppio di quanto già pattuito, e accetterà, in cambio di questo, di chiudere gli occhi sulla sistematica violazione delle libertà democratiche in Turchia e sul massacro del popolo curdo; quello stesso popolo curdo che - come noi ben sappiamo - è stato per molto tempo l'unico avamposto

ma anche del tutto inutile. E anche su questo fronte davvero si imporrebbe un rovesciamento strategico radicale. Lo chiediamo da tempo immemorabile ormai: bisogna aprire subito i corridoi umanitari. Ogni giorno che passa è un giorno drammaticamente dentro questa vicenda. L'Unione deve garantire un sostegno reale e tangibile ai Paesi che costituiscono le frontiere esterne dell'Unione. Abbiamo detto tante volte anche in quest'Aula che è urgente la concessione di permessi di soggiorno per motivi umanitari e che non si può lasciare alla sensibilità dei singoli Governi nazionali la scelta sulla concessione del diritto di ingresso nel loro territorio per i profughi. All'Ungheria, alla Macedonia, alla Slovenia, alla Svezia, alla Danimarca, all'Austria, tutti quei Paesi che fanno della chiusura delle frontiere la sola strategia, andrebbe chiarito che questo equivale davvero a mettersi fuori dall'Europa e dalla civiltà europea, perché significa rifiutare i princìpi costitutivi della identità e della missione che ci siamo voluti dare negli anni passati. Credo che, se l'Europa si muoverà in questa direzione, salverà migliaia di vita e salverà anche il principio irrinunciabile della difesa sempre e comunque della dignità umana, e salverà anche se stessa. Se il presidente Renzi difenderà questi principi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e prossimi mesi, nonostante i profondissimi dissensi che ci dividono da lui sull'operato del suo Governo e nonostante le tante

a prescindere dal fatto che siamo una forza di opposizione, avrà ovviamente tutto il nostro sostegno su un punto come questo. Quando si parla della civiltà

cercando di non ripetere tutte le considerazioni intelligenti - non tutte sono stati intelligenti, ma molte sì - che ho sentito

ciò pone un problema di funzionamento delle istituzioni europee. Come non dargli ragione. Ma io temo che il problema oggi sia diverso: non c'è più solo un evidente problema di funzionamento delle istituzioni. Qui c'è una drammatica crisi dell'Europa; c'è una drammatica caduta di quei valori ideali e di quel disegno politico che i nostri Padri della Patria hanno posto al centro, insieme all'atlantismo, dei dati genetici della nostra Repubblica.

il passaporto passando dall'Italia alla Germania e all'Austria. Allora qui non si tratta più di un problema di funzionamento: è un drammatico problema politico a cui lei può rispondere avendo davanti a sé un bivio. Lei può invocare una strada, che è quella di chi pensa di salvarsi la coscienza dicendo «Noi l'avevamo detto», e lei avrebbe oggettivamente, al di là di qualche amico smemorato che ha parlato prima, prima, qualche carta in regola per dire questo. È da anni, infatti - ad esempio - che diciamo della Turchia le cose che lei ha ricordato. È da anni che diciamo che, se non c'è un controllo esterno delle frontiere, si ricreeranno le frontiere interne. Noi è da anni che diciamo sì agli

L'altra strada che lei ha è assumersi la responsabilità che le compete. Perché qui sta cadendo l'edifico europeo. Lei non può salvarsi la coscienza; lei è un *leader* che

e del mandato che il nostro Parlamento le ha dato: deve cercare di evitare la catastrofe europea, cogestendo con la signora Merkel la ricostruzione dell'Europa. colleghi, i giornali di questi giorni sono pieni della descrizione delle difficoltà della signora Merkel. Io sono angosciato da questo.

nostra. Venendo da quella parte d'Europa, sono angosciato dall'idea che ci siano tanti sciocchi che si compiacciono per le difficoltà della Merkel. Colleghi, le difficoltà della Merkel sono le difficoltà dell'Europa. Se non regge la Germania e se non regge la grande coalizione in Germania, noi andremo alla catastrofe. E noi dobbiamo essere grati alla Cancelliera tedesca, che in questi mesi ha detto ciò che la coscienza europea e i governanti europei non avevano più il coraggio di dire, cioè che l'umanità e i valori costitutivi dell'Europa a volte vengono prima

O i governanti europei cercano di guadagnare qualche voto speculando sulla paura della gente o hanno la capacità di fare ciò che fece Helmut Kohl quando stabilì la parità del marco. Non c'era la parità del marco tra Germania Est ed Ovest e tutti erano contrari, dalla Banca centrale tedesca alle organizzazioni dei lavoratori e dei sindacati confindustriali, ma Kohl stabilì la parità del marco, e così salvò l'unità della Germania e dell'Europa. A me non interessa nulla delle dinamiche che possono portare voi domani a uscire da quella stanza dicendo chi ha ragione e chi ha torto. Io pretendo che il Presidente del Consiglio del mio Paese, se è un *leader* politico che in Europa vuole esprimere la stessa forza travolgente che ha avuto in Italia (a qualcuno fa piacere e a qualcun'altro dispiace: io sono di una generazione che tutto sommato potrebbe trarre non solo dei piaceri da questo evento), deve

Ma oggi si sente, nel rapporto tra Germania e Francia, che manca quella sintonia italiana che deve portare il nostro Presidente del Consiglio a prendere per mano la signora Merkel e, insieme, l'asse del Partito socialista europeo e quello del Partito popolare europeo nella ricostruzione dell'Europa. Se cade Schengen, cade l'Europa. Noi dobbiamo confrontarci con una realtà di egoismo della quale abbiamo responsabilità anche noi. Quante volte abbiamo detto, davanti a scelte impopolari, noi dirigenti politici dei nostri Paesi, che facevamo quella riforma perché lo chiedeva l'Europa.

Sono contento che il Presidente del Consiglio del mio Paese abbia detto che quest'accordo non ci deve obbligare a vendere l'anima e credo che la sua dichiarazione dopo lo scorso Consiglio europeo abbia fatto fatto sobbalzare positivamente molti, perché sembrava veramente che andassimo ai saldi di fine stagione. Dopodiché, abbiamo bisogno della Turchia almeno quanto la Turchia ha bisogno di noi. Per cui, alla fine diamo la partita in pareggio. porre con forza la questione del Mediterraneo. Quante volte abbiamo detto che senza una politica del Mediterraneo sarebbero venuti solo guai? E, infatti, è così. Tutti i guai ci stanno venendo dal Mediterraneo. Ritengo ottimo, ad esempio, che il Presidente della Repubblica in questo momento sia in Africa, come ritengo positivo che ci sia andato lei perché questo significa che capiamo la realtà. Quando un continente naviga tra al-Shabaab, Boko Haram e al-Qaeda in competizione con l'ISIS e tutti nell'Africa spingono su questo flusso di disperati verso le nostre coste, è chiaro che se noi non pacifichiamo l'Africa avremo un Mediterraneo in fiamme e non riusciremo a fare nulla per evitarlo. Il senso Il senso del mio accorato intervento è allora questo: crediamo che il Governo italiano - certo, l'Italia non è una superpotenza, ma è uno dei grandi Paesi europei ed è uno dei Paesi fondatori il Governo del nostro Paese è più forte di molti altri Governi - deve dare una mano, soprattutto in direzione di un rapporto rinnovato tra Italia e Germania, a chi si propone di essere l'alternativa allo sfascio dell'Europa. Quando avremo sfasciato l'Europa, tanti che scioccamente hanno fatto il verso capiranno che chi è più penalizzato da questa prospettiva è proprio l'asse mediterraneo e il nostro Paese in primo piano. Noi oggi difendiamo ideali che coincidono con i nostri interessi e vogliamo che il nostro Governo lo faccia con rinnovato supporto del Parlamento.

che il nostro Presidente del Consiglio può benissimo accelerarla e aiutarci a fare chiarezza su questi delitti di Stato e non certo di terrorismo islamico, che dovrebbe essere l'oggetto di questo Consiglio europeo. Ancora una volta ci troviamo ad affrontare due temi di cui spesso si parla nel Consiglio europeo: la crisi economica e quella migratoria. Il motivo per cui si parla sempre di queste cose è perché le soluzioni trovate in Europa e dai Governi sono del tutto insoddisfacenti. cosa per chi ci ha accusato di voler mettere reti e fili spinati, mentre per noi nessuno deve rimanere indietro, pertanto, non ci nominate quando parlate di razzismo voi, che avete fatto i soldi sugli immigrati come se si la crisi migratoria ha portato alla luce il collasso morale dell'Europa. Vi ricordo che l'Unione europea conta più di 500 milioni di abitanti e nel 2015 abbiamo accolto soltanto 1.200.000 richiedenti asilo. Si tratta per questa Unione europea che dovrebbe essere la culla della solidarietà. Per questi numeri esigui abbiamo assistito a Governi che hanno richiesto l'abolizione di regole e principi fondanti l'Unione europea,

tutto rinviato a questo incontro, e mi sarebbe piaciuto sentire il presidente Renzi parlare di quello che ha intenzione di dire e non di lutti, mafia e delitti di Stato. Però, pazienza, questo è quello che offre la casa: nessuno lo ha eletto all'accordo sull'immigrazione che ci si appresta a siglare nella prossima riunione del Consiglio europeo, mi sembra che l'unica cosa intellegibile detta dal *premier* Renzi durante il suo intervento è che dirà sì al ricatto della Turchia. Ciò è gravissimo, perché l'accordo che ci si appresta a siglare è per fare un patto del diavolo con la Turchia. Mai come oggi la Turchia è lontana dai principi democratici che dovrebbero ispirare la nostra Europa. Quello che ci apprestiamo a fare è delegare il lavoro sporco - un siriano per un siriano - a un Paese come la Turchia che, mai come adesso, è stata lontana dai principi democratici che ispirano l'Unione europea e sta ricattando l'Europa, che si trova in ginocchio.

la Turchia è un alleato infedele, come dimostrano le ripetute violazioni dell'accordo doganale con l'Unione europea, il blocco alle frontiere di TIR e merci europee, l'aumento ingiustificato dei dazi doganali, la chiusura delle imprese italiane e la politica protezionistica praticata dal Governo. Erdogan pretende, ma non stringe la mano tesa e usa i rifugiati per ottenere i soldi europei, mentre Libano e Giordania non ricattano nessuno e ospitano milioni di rifugiati in più rispetto alla Turchia.

siamo noi che abbiamo creato questo disastro e l'unica cosa intelligente che si può fare è stabilire l'embargo delle armi all'Arabia Saudita, in modo che si rispetti veramente la dignità di questi popoli, impedendogli di essere uccisi dalle nostre armi.

ci rimprovera quando, trattandosi un qualsiasi argomento, noi andiamo fuori tema. Oggi però non l'ha interrotta; lei doveva parlarci del Consiglio d'Europa e invece ci ha parlato di tutt'altro. Ci ha parlato di politica interna, di economia e di infrastrutture, tutte cose assolutamente importanti, ma assolutamente fuori tema. Quindi io la prego, signor presidente Grasso, utilizzi lo stesso trattamento per tutti i componenti di quest'Aula e per tutti i rappresentanti del Governo. Governo. Noi non abbiamo appreso nulla di ciò che il nostro Governo si appresta a fare nel prossimo Consiglio d'Europa. È una ritualità il Consiglio d'Europa ed è anche una ritualità questo incontro che noi facciamo? Rivediamo allora i nostri calendari, perché credo che questo possa essere importante. Due piccolissimi spunti voglio darle, signor Presidente del Consiglio, dato che va a difendere e a discutere degli interessi dell'Europa, ma, all'interno di quegli interessi, va a difendere gli interessi italiani.

non può essere fatta sulla pelle degli agricoltori italiani, e meridionali in particolare. Dato che stiamo parlando delle cose più varie, perché non si parla di Europa, allora parliamo principalmente di questo. Questa decisione assunta dalla Commissione europea incide profondamente sugli interessi della nostra agricoltura. Potrei citare cento e tanti altri casi di distrazione del Governo italiano, nel momento in cui va a discutere dei problemi essenziali dell'economia del nostro Paese in Europa.

interventi strutturali, per poter agevolare quella decontribuzione (che non è fiscale, ma è previdenziale) sulle nuove assunzioni, che oggi le ha consentito di citare qualche cifra, ma che fra tre anni ci porterà porterà sul groppone gli esiti di una bolla occupazionale, dato che quelle previsioni di assunzione agevolata non sono collegate a nessun meccanismo di stabilizzazione degli stessi posti di lavoro. Quindi possiamo parlare di tutto e di più. Oggi poi il tempo è brevissimo. Io spero che comunque nella prossima riunione lei affronti dal punto di vista delle migrazioni, dato che affronta il tema di un ulteriore finanziamento alla Turchia, il quesito non risolto della clausola migranti, sono stati impegnati da noi parecchi denari; lei ha utilizzato una parte di quegli impegni per poter finanziare alcune attività previste dalla legge di stabilità. Che fine ha fatto la clausola migranti? Che fine ha fatto l'ultima nota che l'Unione europea ci ha inviato riguardo alla legge di stabilità dello scorso anno? Abbiamo chiesto che il Ministro dell'economia venga a riferire con urgenza in Commissione bilancio su questi avvenimenti. Sono tutti argomenti certamente di grandissimo rilievo, che però qua non sono stati neanche sfiorati. Abbiamo sentito di una serie di cose fatte, a nostro giudizio maldestramente e a suo giudizio positivamente, ma non abbiamo sentito parlare

Devo chiudere. La ringrazio, signor Presidente del Consiglio, e spero che questo dibattito sulle cose interne possa essere affrontato nella sede competente, quindi con il preannuncio dovuto secondo il nostro calendario. desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, per la sua comunicazione. La questione migratoria rappresenta per l'Italia e per l'Unione europea una grande minaccia e, al tempo stesso, una grande opportunità. La minaccia è quella di consentire alle forze politiche che hanno un progetto contrario e opposto a una più forte integrazione degli Stati membri di approfittare e strumentalizzare una grande tragedia umanitaria dalle dimensioni planetarie, per attaccare, corrodere, disgregare, spezzettare le istituzioni europee, far crescere nuovi steccati, erigere muri e filo spinato e, soprattutto, reintrodurre barriere commerciali, ostacoli al libero scambio delle merci e alla libera circolazione delle persone, riattivare politiche economiche protezionistiche e barriere doganali, nella convinzione che dalla crisi si possa uscire meglio da soli, magari ripristinando una valuta nazionale e facendo leva sulla scorciatoia di una svalutazione, come ai tempi della lira. In altre parole, si vuole tentare la strada della competizione internazionale non attraverso la solidità di un impianto produttivo, della qualità intrinseca delle merci e dei prodotti che produciamo, dell'efficienza dell'apparato amministrativo e giudiziario, ma attraverso la politica "dopata" della svalutazione artificiosa della moneta e, dunque, dei prezzi. Questo è il vero obiettivo politico che viene perseguito dalle forze antieuropeiste, che non a caso sono le stesse che oggi si oppongono, con argomenti fondati sulla paura e sul risentimento, a qualunque politica che miri a regolare i flussi migratori. Per loro vale il detto «tanto peggio, tanto meglio», in quanto appaiono loro chiari i dividendi a breve termine di una speculazione politica, che consente di lucrare consenso, facendo leva proprio sui sentimenti di smarrimento e di legittima e di legittima preoccupazione, che sentono tanti nostri connazionali, di fronte ad una tragedia umanitaria di così vaste proporzioni. Non stupisce che siano le stesse forze politiche che negli anni passati, governando da destra le istituzioni dell'Unione europea, ne abbiano indebolito la capacità di reazione, ne abbiano favorito la sclerosi burocratica, ne abbiano ridotto all'osso il bilancio; in altre parole ne abbiano favorito e persino determinato l'apparente paralisi decisionale e la miopia sulla visione strategica da adottare, per affrontare una situazione così complessa, come quella delle migrazioni e dei disequilibri macroeconomici tra le diverse aree del Nord e del Sud del mondo. Il calcolo di queste forze politiche, che come abbiamo visto anche oggi affidano la loro propaganda soprattutto all'insulto, al dileggio, all'offesa personale, ad espressioni truci e volgari, è un calcolo miope, che danneggia gli interessi del nostro Paese. Esse si rendono alleate, non so fino a che punto consapevoli, di quelle forze politiche e finanziarie, ben collocate in alcuni distretti industriali nordeuropei, che vorrebbero assegnare ai Paesi della sponda mediterranea, come l'Italia, la Spagna e la Grecia e alcuni Paesi balcanici, una mera funzione di filtro, un vasto territorio destinato semplicemente a trattenere e disperdere le ondate di migranti provenienti dai Paesi del Maghreb e del Nord Africa. In altre parole, si vuole trasformare l'Italia, che verrebbe ovviamente esclusa dalle zone euro e Schengen, in una specie di Turchia o di Libia; insomma in una zona cuscinetto, atta a proteggere le ben funzionanti e ricche economie dei Paesi nordeuropei. Questo progetto politico, nemmeno tanto velatamente propugnato da forze che, anche a causa della debolezza e inanità di nostri precedenti Governi, in tutt'altre faccende affaccendati, hanno metodicamente preso il controllo di tutte le leve di controllo e di governo delle istituzioni europee, oggi trova inaspettato appoggio in quelle forze politiche nazionali, che non essendo riuscite a dividere l'Italia, vorrebbero dividere l'Europa; una specie di quinta colonna, gli utili sciocchi che volentieri si prestano ad aiutarle a fare del nostro Paese una realtà politica insignificante e marginale. Se dunque oggi ci opponiamo a questa politica che vuole disgregare l'Europa, che intende strumentalizzare la tragedia dei migranti per disarticolare le istituzioni europee e reintrodurre le frontiere, non è per ingenuo buonismo, ma perché siamo profondamente convinti che il rafforzamento dell'Unione europea e l'attribuzione ad essa di un ruolo centrale nella politica migratoria corrisponda ad un rafforzamento degli interessi nazionali e dei nostri concittadini. Siamo noi che intendiamo difendere gli italiani, con politiche serie e di lungo raggio e non a colpi di *slogan* ad effetto più o meno truculenti. Come dicevo, signor Presidente, la questione migratoria è una grave minaccia, ma anche una grande opportunità per l'Italia e l'Unione europea: quella di dimostrare la perdurante vitalità e forza dei valori sui quali esse sono state fondate e sono cresciute, valori che hanno consentito non solo il più lungo periodo di pace di cui abbia mai beneficiato nella sua storia il nostro continente, ma anche il più alto livello di sviluppo economico mai raggiunto. Oggi vediamo con un certo sgomento verificarsi la profezia di Albert Camus che, parlando metaforicamente della peste ma alludendo all'intolleranza e alla violenza, infatti, quello che ignorava la folla e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere e che forse sarebbe venuto il giorno in cui la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice». L'Europa è stata per molto tempo questa città felice e noi non possiamo permettere che i bacilli del razzismo, dell'intolleranza, della xenofobia, della segregazione, della discriminazione tornino a insudiciare il nostro continente. Segnali preoccupanti giungono anche dai risultati elettorali dei giorni e delle settimane scorse ed è necessario che chiunque abbia animo democratico e amore per la libertà sia vigilante. L'Italia e l'Europa devono essere all'altezza dei loro valori fondativi: unità nella diversità è il motto europeo; sono parole scritte con il sudore e con il sangue di tanti cittadini europei che si sono dovuti mettere in cammino e attraversare frontiere in cerca di una esistenza migliore: penso ad esempio ai morti di Marcinelle, dove sessant'anni fa morirono 262 minatori in gran parte italiani. Dovremmo ricominciare da quella memoria per ritrovare il senso del nostro futuro. L'Europa deve dotarsi non solo di una politica per l'immediato, ma sviluppare una strategia di più ampio respiro, mirata non solo a contenere o regolare l'ondata migratoria ma a normalizzare e governarne i flussi. Occorre innanzitutto abbandonare l'impostazione della legge Bossi-Fini che rende qualunque migrante un clandestino: come si può oggi entrare legalmente in Italia? È praticamente impossibile ed è dunque da ipocriti distinguere tra chi è presente legalmente e chi è clandestino perché è la legge stessa a rendere tutti clandestini. Soprattutto è necessario ridurre gli enormi squilibri macroeconomici tra le diverse aree del mondo. Nei mesi scorsi a Malta, nel corso del *summit* a La Valletta, l'Unione europea ha stretto accordi con i Paesi africani da cui fugge o transita la maggior parte dei migranti che dal Continente nero si dirigono verso l'Europa. Con questo accordo si è voluto compiere un salto di qualità importantissimo nelle relazioni con gli Stati dell'Africa sub-sahariana per una cooperazione rafforzata e più efficace nella lotta contro l'emigrazione irregolare e la tratta di persone nel Mediterraneo. Si sta tentando di creare una sorta di cintura di sicurezza sulle rotte dei Paesi di origine e di transito dei flussi migratori che hanno come destinazione l'Europa: la Horn of Africa migration route, ovvero Djibouti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Tunisia. Forse proprio su questo fronte converrebbe concentrare sforzi e impegno, piuttosto che insistere esclusivamente sull'accordo con la Turchia. Il processo di Khartoum, di cui l'Italia ha sin dall'inizio avuto la regia, oltre a fornire il quadro di riferimento che mancava per una politica strutturata ed un confronto operativo tra l'Unione europea ed i Paesi del Corno d'Africa, ha strutturato un percorso ambizioso teso ad affrontare le cause profonde dell'immigrazione di massa, evidenziando lo stretto legame tra quest'ultima e l'assenza di prospettive di sviluppo. Di fatto la EU-Horn of Africa migration route initiative si propone di controllare questi flussi attraverso intese che prevedono piena collaborazione dagli Stati africani a fronte di investimenti in cooperazione. Qui però c'è un punto dolente. Governi, o meglio regimi, che sono ritenuti inaffidabili dalle organizzazioni non governative per i diritti umani e che, nonostante il supporto - anche economico - dell'Unione europea, non sono riusciti a mettere in atto processi di democratizzazione e di inclusione sociale al proprio interno, possono davvero fermare i flussi migratori? Quali garanzie possono fornire sul rispetto dei diritti dei profughi e su eventuali forme di corruzione nella gestione dei campi? In conclusione, è necessario prevedere forme di monitoraggio per assicurarsi che gli accordi vengano di fatto rispettati e al tempo stesso operare affinché essi evolvano verso pratiche più rispettose dei fondamentali diritti civili e democratici di quei popoli; un'impresa difficile che solo l'Europa unita può conseguire. signor Presidente, mi lasci dire che proprio questa mattina i giornali hanno pubblicato un documento che è stato ritrovato nel quattrocentesimo anniversario della morte di William Shakespeare, il più grande

Che sia in Francia o Fiandra, in qualsiasi provincia germanica, in Spagna o Portogallo, anzi, ovunque non rassomigli all'Inghilterra, orbene, vi troverete per forza a essere degli stranieri. Vi piacerebbe allora trovare una nazione d'indole cosi barbara che, in un'esplosione di violenza e di odio, non vi conceda un posto sulla terra, affili i suoi detestabili coltelli contro le vostre gole, vi scacciasse come cani, quasi non foste figli e opera di Dio, o che gli elementi non siano tutti appropriati al vostro benessere, ma appartenessero solo a loro? Che ne pensereste di essere trattati così? Questo è ciò che provano gli stranieri. Questa è la vostra disumanità».

Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli senatrici, il dibattito è stato ricco, con tredici interventi. L'ho seguito con attenzione e vi ringrazio per gli stimoli che avete portato e che spero di poter consegnare alla discussione di domani e di venerdì. Ringrazio tutti e, da ultimo, il senatore Cociancich per la sua citazione di Shakespeare. Ieri tutti noi siamo rimasti molto colpiti da un'immagine che ritraeva l'attraversamento di un fiume, dove peraltro tre persone hanno perso la vita.

Giovanni Paolo II proclamò il patrono dei politici, naturalmente per i cattolici che fanno parte di questo consesso), mi hanno fatto pensare e quindi la ringrazio per le sue considerazioni. interpreterei il mio concetto di replica offrendo alcuni dati all'attenzione dei senatori che sono intervenuti, anche con un eccesso - se vorrete - di pignoleria e di dettaglio, e poi mi limiterei ad una conclusione politica sulla base delle considerazioni che diversi hanno svolto e tra questi, in modo particolare, il senatore Casini. Parto dalle questioni che ha sollevato la senatrice Lezzi. Anch'io mi unisco al bentornato, in queste ore, alla senatrice, e affido la mia replica ai suoi colleghi immaginando che abbia degli impegni comprensibili in questo caso. La senatrice Lezzi ha sollevato una polemica che io non condivido sui numeri del Governo italiano. Vorrei semplicemente citarne alcuni perché ciascuno si faccia la sua opinione e perché chi vuole possa poi passare al *fact checking*, cioè il controllo dei dati reali.

Ho grande stima del dottor Marchionne e, a differenza di altri, presenti anche in questa sala e anche nella mia parte politica, lo ritengo un punto di riferimento molto importante per l'economia italiana; se ci sono dei timidi segnali di ripresa, questo deriva anche dal fatto che siamo tornati a fabbricare auto in Italia e che in Basilicata si fabbrica una vettura della Jeep per gli Stati Uniti. Ma messa a fattor comune questa grande stima che nutro nei confronti del dottor Marchionne, mi sento di escludere che il suo stipendio stia sotto i 1.500 euro netti al mese. I dieci milioni di italiani che prendono gli ottanta euro, per i quali tutto è tranne che una mancetta come spregiativamente alcuni politici lontani dalla realtà tendono a definire questa misura, hanno con gli ottanta euro la possibilità di uno spazio di vita quotidiana decisamente importante e significativo. Io non voglio convincervi della bontà della strategia economica di questo Governo, ma spero che dopo due anni e un mese di azione sia chiaro che gli ottanta euro non sono un *bonus* elettorale. Aggiungo - giusto per raccontare la realtà per com'è - che ce lo siamo dimenticati, ma gli ottanta euro sono arrivati dopo le elezioni europee, perché essendo pagati il Immagino cosa possa concepire un italiano a casa: c'è un Governo che sta abbassando le tasse e gli altri che discutono se le ha abbassate il giorno prima o il giorno dopo le elezioni. Sono due anni che dieci milioni di italiani,

La cosa più straordinaria è che più fanno polemica autorevoli esponenti... che fanno più polemica autorevoli esponenti di Governi che furono, che adesso si lamentano di noi per questa misura; se è una misura così importante perché

per l'aspetto comunicativo ci sarà qualcuno che dice, da parte del Governo, che abbiamo ridotto le tasse a dieci milioni di italiani, e il senatore Scilipoti Isgrò che dice che non è giusto dare ottanta euro a dieci milioni di italiani che non arrivano a 1.500 euro al mese.

Vorrei che fosse chiaro, per la senatrice Lezzi e per tutti noi, che il dato del PIL, su cui si è a lungo discusso perché era previsto lo 0,7, poi lo 0,9 e si è chiuso a 0,8 (e ciò ha aperto una grande discussione), è il primo dato positivo dopo tre anni di segno meno. Ora uno più discutere: «Però mi aspettavo di più: io avrei voluto prendere l'1,5 perché perché gli altri hanno fatto 1,5, 1,3, 1,0,5, 1,7...»; tutte cose assolutamente sacrosante, ma il dato di fatto è che l'Italia viene da un triennio di segno meno,

Io penso che se l'Italia avesse fatto, tra il 2003 e il 2005, quello che ha fatto la Germania, cioè una riforma del mercato del lavoro, per il nostro Paese sarebbe stato meglio, e lo dico senza aprire una discussione polemica, ma prendendo atto del fatto che la Germania nel 2003 ha iniziato con Schroeder una riforma del mercato del lavoro che ha chiuso nel 2005 con la Merkel. Non vi è stato uno scontro su questo. Fatto sta che oggi il tasso

Cito sia il dato ISTAT dalla disoccupazione sia i numeri del *jobs act*, perché credo che su questo vada lasciata agli atti di questo Senato la realtà per quella che è.

ma non c'è ombra di dubbio rispetto al fatto che passare dal 13 all'11 per cento - credo che almeno su questo converrà persino il senatore Scilipoti Isgrò - è segno di un miglioramento.

perché si può essere d'accordo o in disaccordo su tutto, ma non si può fare a cazzotti con la realtà. Vorrei citare i dati dell'INPS e dell'ISTAT.

- delle assunzioni e delle trasformazioni, con il segno meno delle cessioni (poi arrivo anche alle persone, non ho fretta). Il punto centrale, dunque, è che almeno si possa mantenere un minimo di realtà; poi si ragiona di politica e si fa la discussione che il senatore Casini ci ha opportunamente sollecitato. Ma il dato di fatto è che, ad oggi, i dati INPS segnano in Italia - e penso che ne siamo tutti contenti, perché credo che nessuno di noi sia insoddisfatto se vi è un contratto di lavoro a tempo indeterminato in più 913.000 contratti a tempo indeterminato. Possiamo dire che vi sono 913.000 persone in più a lavorare? No. E vengo ai dati dell'ISTAT, che si dividono in due categorie: gli occupati permanenti in più e gli occupati totali (così rispondiamo alla considerazione della senatrice Lezzi, che parla di trasformazioni, dicendo che sono tutte trasformazioni). Aprirei volentieri con voi una discussione sul fatto che, se esistono delle trasformazioni, vuol dire che uno che era precario prende il contratto a tempo indeterminato. Certo, a tutele crescenti, che significa a tempo indeterminato perché è un contratto a tutele crescenti. Credo che non si sia iscritto in replica il senatore Ichino, altrimenti potrebbe ampiamente illustrarvi la valutazione su questo istituto giuridico. Il punto, però, qual è? Se io sono un precario, che non ha un contratto a tempo indeterminato, e quindi sono un occupato precario e divento un occupato a tempo indeterminato, forse per voi è solo una trasformazione,

Arrivo al punto: quanti sono gli occupati totali? Quando dico che ci sono 468.000 occupati permanenti in più sto spiegando che esiste un numero che contempla e comprende le trasformazioni di cui la Lezzi ha parlato. Non sto negando che una parte di questi contratti in più siano trasformazioni; ma, a differenza della senatrice Lezzi e dei senatori che urlano del Movimento 5 Stelle, sono convinto che sia comunque un fatto positivo. Ma riconosco che una parte di questi è è semplicemente trasformazione. Cosa dice l'ISTAT (e ho concluso sulla questione del lavoro)? Gli occupati totali in più nel 2015 sono 221.000.

Questo è il risultato del *jobs act*. Poi uno può dire che la parte del *jobs act* normativa incide più o meno rispetto alla parte normativa

Il senatore D'Alì diceva che sono contributi, esoneri di natura previdenziale. Vero, ma sono stati resi possibili dall'eliminazione della componente «costo lavoro dell'IRAP».

Questa parte ha prodotto un risultato totale in Italia di 913.000 contratti a tempo indeterminato in più, 468.000 occupati permanenti e 221.000 occupati in più. Questo cosa significa? Significa che questa operazione ha funzionato. Dite che è stato un colpo di fortuna? Ditelo. Dite che è stato il destino cinico e baro che a voi non l'ha permesso di fare e a noi sì? Io da italiano dico che se questa cosa l'aveste fatta voi dieci anni fa, sarei stato più contento che non venire qui a fare la parte di quello che deve rivendicare al Governo questo risultato. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E sono convinto che la pensino così anche molti vostri elettori e anche molti vostri senatori che, anche per questo, hanno qualche difficoltà rispetto all'attuale situazione della destra.

rapidamente all'ultimo punto. Bisogna che lo faccia perché è un tormentone: «Renzi non sei stato eletto». Alla fine, dopo due anni e un mese, bisogna che citi testo. Poiché ci sono alcuni che vogliono difendere la Costituzione da questi che la vogliono cambiare, da questi pericolosi rivoluzionari - che peraltro non vogliono cambiare questa parte - vorrei citare brevemente l'articolo 92 e l'articolo 94 della Costituzione, con particolare dedica ai senatori Tosato e Marin. comma: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri». Vorrei svelare questo segreto: non è una norma *ad personam*, come quelle che votavate in passato. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questa è proprio una norma che è sempre valsa per gli ultimi 63 Governi e per i 27 Presidenti del Consiglio di questo Paese, quindi non c'è stato nessuno che è stato eletto direttamente. Poi c'è stato chi voleva portare l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non è stata portata avanti per mille motivi, nonostante varie Commissioni bicamerali, e che non fa parte nemmeno del disegno di legge di riforma costituzionale che ci accingiamo a votare in sesta lettura alla Camera. Rispetto Rispetto al giudizio di legittimità che il Presidente del Consiglio deve esprimere o meno, leggo l'articolo 94: «Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere». Senza il consenso di Tosato, che non era ancora senatore perché non era stato eletto, ma questo nulla toglie rispetto alla sua legittimità; cioè, lui non ce l'aveva fatta ad essere eletto, poi si è dimesso il senatore Bitonci ed è entrato lui, ma vale comunque, è un senatore come tutti gli altri, non è un senatore diverso... *(Commenti del senatore Scilipoti

Non l'hanno fatto, però, purtroppo per loro, la Camera e il Senato hanno votato la fiducia a questo Governo. Cosa dice l'articolo 94, Senatore Di Maggio, non può intervenire. La richiamo all'ordine.

Il senatore Di Maggio ha detto «cialtrone» a chi ha scritto questo articolo della Costituzione. Prendo le distanze dalla frase del senatore. Dunque, cosa accade? Accade che nel momento in cui il Governo mette la fiducia e non la ottiene, il Governo va a casa. Ora, si può dire tutto al nostro Governo, ma non che non abbiamo messo tante volte - arrivo a dire forse un po' troppo - la questione di fiducia in quest'Assemblea; e tuttavia la fiducia ci viene confermata tutte le volte. Questo vuol dire che, nonostante abbiamo avuto 54 tentativi, questo Governo è legittimo, la Costituzione è salva, la vostra incapacità di leggere i fatti giuridici di questo Paese è impressionante.

però questo giudizio di natura costituzionale si scontra con la realtà dei fatti. In realtà, è accaduto un fatto clamoroso alle ultime elezioni europee,

dei ministri*. È impressionante come non si rendano conto di fare il gioco degli altri. È proprio una cosa imbarazzante. Il punto centrale, senatore Di Maggio, è che da qualche decennio in questo Paese i voti si considerano sulla base della percentuale che viene raggiunta da ciascun partito. Quel partito ha preso il 40,8 per cento. Accettiamo, però, la proposta del senatore Di Maggio e guardiamo i voti assoluti.

con 10,6 milioni di voti. Quindi, i due partiti più votati sono stati il Partito Democratico italiano, nonostante il mancato appoggio del senatore Di Maggio, e il partito della cancelliera Merkel.

il bivio è molto semplice: o noi, tirandoci su le maniche, cerchiamo di recuperare e di ricostruire un'idea d'Europa che abbia i valori che cinquantotto anni fa hanno segnato la storia di Roma, e non soltanto di Roma; oppure stiamo andando a sbattere in quei tornanti della storia che un grande cristiano democratico italiano usava definire come momento chiave dell'esperienza politica e che sono tornanti della storia di rara pericolosità. Intorno alle questioni dell'immigrazione, della crescita, della sicurezza e securitaria sono soltanto la conclusione e le parole di un documento del Consiglio europeo, e c'è l'idea stessa di ciò che ha portato i Padri fondatori a immaginare l'Europa.

certi legittimi sentimenti di rabbia, il nostro sforzo è esattamente in questa direzione: fare di questa stagione, non una stagione di polemiche interne e di egoismi, ma una stagione costituente e ricostituente per l'Europa, perché l'Europa dei figli sia all'altezza del sogno dell'Europa dei Padri.

verrebbe così riformulato: «a sostenere l'attuazione di una dimensione sociale dell'Unione europea, inclusi strumenti comuni di garanzia contro la disoccupazione». Nel paragrafo successivo si propone di sostituire «a rifiutare il piano Schauble» con «a rifiutare qualsiasi piano».

se così riformulati: nel primo, anziché «sollecitare», a «ribadire la necessità di attuare gli accordi relativi alla gestione dei flussi migratori» e il resto viene mantenuto; nel secondo impegno sostituire «richiedere» con

risoluzione n. 6 il parere è contrario alle premesse e favorevole agli impegni, se vengono accettate le riformulazioni del Governo

tutti i senatori presenti in Aula e che, quindi, non conosca l'anonimo senatore Tosato. Sappia, comunque, che quando sono stato eletto in Senato ricoprivo la carica elettiva di consigliere regionale. Facevo parte di quella categoria di rappresentanti dei cittadini che oggi il Presidente del Consiglio vorrebbe portare in massa in Senato. Potrei dire, ma non lo penso, che sono il miglior prototipo del senatore che Renzi vorrebbe in quest'Assemblea. Il Presidente del Consiglio deve poi rendersi conto di un'altra questione.

ma credo che sia veramente triste che un Presidente del Consiglio non abbia l'autorevolezza di rispondere alle osservazioni politiche dei senatori di quest'Assemblea, trasformando il dibattito in una questione personale. Noi non abbiamo bisogno di un fenomeno o di uno spaccone al Governo, avremmo semplicemente bisogno di un Presidente del Consiglio che abbia a cuore la vita dei cittadini italiani. Purtroppo, in questo momento l'Italia non ha questo Presidente del Consiglio.

poche brevi parole. Sono state molto sagge le parole del presidente della Commissione affari esteri, il collega Casini: il problema dell'Unione europea e il problema del Governo italiano è un problema di mancanza di *leadership*. La mancanza di *leadership* da cosa si vede? Da un fatto semplicissimo. È stata posta una domanda molto concreta: ha ragione il ministro Alfano quando dice che non c'è alcun rischio sulla cosiddetta rotta adriatica e che mai nessuno arriverà in Italia dall'Albania, ha ragione il comandante del contingente KFOR NATO a Pristina, che dice invece che le truppe NATO sono state allertate perché occorre trasportare in Albania decine di migliaia di persone provenienti dalla Turchia? È una questione semplice; bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome e di rispondere alle domande. Altrimenti cosa accadrà? Domani Renzi andrà a Bruxelles, siederà a quel tavolo, ovviamente non potrà dare alcuna risposta, ma soprattutto sarà inconsapevole rispetto ai contorni di un accordo Unione europea-Turchia che lascia aperta la possibilità di scatenare la rotta adriatica. Quindi, con un Governo che ammette di partecipare ad una riunione di inconcludenti, non c'è forse il rischio che, tra quelli seduti al tavolo, il più inconcludente di tutti sia esattamente quello che soccombe?

che il Governo ha accettato con delle riformulazioni, abbiamo illustrato nel dettaglio le ragioni che ci spingono a sollecitare un'azione più decisa del Governo in sede comunitaria. Da questo punto di vista il prossimo Consiglio europeo, anche al di là dei risultati immediati che si potranno ottenere, rappresenta un'occasione importante che non può essere mancata. Di fronte a quel consesso è necessario che l'Italia parli il linguaggio dell'Europa, ma di un'Europa diversa da quella che siamo abituati a leggere nelle cronache giornaliere; di un'Europa aperta e aperta e rispettosa degli obblighi internazionali, ma anche rigorosa nel difendere i propri cittadini da possibili invasioni, che, per quanto umanamente comprensibili, si scontrano tuttavia con la logica dei grandi numeri. Il fenomeno dell'immigrazione, tipico dell'epoca moderna ed esso stesso figlio della globalizzazione, non può essere ignorato, ma non può nemmeno non essere gestito avendo come bussola ed orientamento quelle regole che che rappresentano il nostro vissuto quotidiano. Occorre, per quanto possibile, un contingentamento e una gradualità, in cui il conto delle risorse a disposizione e dei bisogni da soddisfare abbia una base razionale. Cedere all'impulso del momento, com'è avvenuto in altri Paesi, non fa altro che alimentare il malessere sociale e quei fenomeni di becero populismo che rischiano di avere effetti perniciosi per l'intera stabilità politica dell'Europa, che ha bisogno di ritrovare tutta la sua originaria ispirazione comunitaria, invece di rinchiudersi nel recinto dei propri confini. In un momento di emergenza come quello attuale, la cosa peggiore sarebbe cedere ad impulsi irrazionali, anche se rivestiti dall'etica della solidarietà, per poi scatenare reazioni xenofobe, che riportano indietro le lancette della storia. Se questo vale per la Siria, dove tuttavia si è accesa una piccola fiammella di speranza a seguito del ritiro delle truppe russe, per la Libia la situazione è ancora più preoccupante. Lo dico con prudenza: nessuna avventura. In passato abbiamo già dato ed è stato un errore; perseverare sarebbe addirittura diabolico. Lasciamo quindi ad altri i propositi guerrafondai. Ogni intervento militare, per quanto ci riguarda, come Gruppo, non può che che essere la conseguenza di una richiesta da parte del Governo libico ed avere tutti gli *imprimatur* di carattere internazionale. Intervenire fuori tempo sarebbe solo la rinnovata certificazione di una vocazione neoimperialista, che l'Italia, visti i suoi trascorsi storici nella Regione, non può permettersi. Quindi calma, colleghi. Riflettete sulle parole che sono «dal sen fuggite» allo stesso Barack Obama, nella sua critica puntuale all'operato di Cameron e di Sarkozy. ben più fermo di quanto, a suo tempo, fece Silvio Berlusconi, attratto, seppure a malincuore, visto la sua critica postuma, dalle sirene francesi ed inglesi.

quale lotta contro i suoi potenti oppositori interni al *board* e deve subire i continui attacchi della stampa benpensante tedesca. Dall'altro c'è la Commissione europea, che rema in una direzione opposta e contraria, che insiste su politiche di rigore, che hanno senso quando l'inflazione l'inflazione mina le basi della credibilità finanziaria, ma che ottengono effetti contrari quando l'orizzonte è quello della deflazione. La verità è che la BCE e la Commissione europea perseguono politiche contrapposte. La prima tenta di portare l'inflazione al 2 per cento per rilanciare l'economia reale e la seconda la gela, con regole di bilancio, all'insegna dell'austerità e del contenimento finanziario. Essa non deve essere necessariamente spesa corrente e cibo per cicale, ma può essere rilancio degli investimenti, tanto più efficaci, se accompagnati da riforme in grado di rimettere in moto il mercato. Invece si procede in direzioni contrapposte, segno che la Commissione europea non ritiene valido l'obiettivo di un 2 per cento del tasso d'inflazione. Ma è la Commissione che può decidere questo o non spetta al Consiglio europeo stabilire quale sia la rotta da seguire? Questo dualismo va quindi risolto nel più breve tempo possibile. Se si ritiene che Draghi sbaglia, allora - cosa improbabile e estremamente pericolosa per le sorti stesse dell'Europa - si cambi il vertice della BCE. Se però Draghi, come ritengo, ha ragione, allora è il Consiglio europeo che deva battere un colpo, tracciare la strada da seguire, casomai dopo averne discusso nel Parlamento europeo, indicare obiettivi vincolanti, all'interno dei quali far muovere la successiva attività della

Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, questo vertice arriva in un momento molto difficile, con gli attentati dello scorso fine settimana, la Siria, l'evolversi della situazione libica e, purtroppo, l'incapacità delle organizzazioni sovranazionali a far fronte a queste emergenze. Ieri ricorreva il quinto anniversario dall'inizio della guerra in Siria: sono morte 450.000 persone, sono milioni gli sfollati e altrettanti quelli che sono pronti a lasciare il Paese. C'è poi un dramma nel dramma ed è quello dei bambini che in questi cinque anni non hanno mai messo piede in una scuola, sono orfani e apolidi, perché nati nei campi profughi. Le polizie internazionali calcolano che nel nostro Paese ci siano circa 5.000 minori di cui non si ha più notizia. Davanti a eventi di una così grande portata, ci vuole il massimo sforzo dell'Unione europea. Lo abbiamo detto più volte in quest'Aula e più volte lo ha detto lei, lo ha detto il Presidente del Consiglio, qui come nei consessi internazionali. Tuttavia è evidente che, nonostante la buona volontà di Paesi come il nostro, l'Europa mostra ritardi e contraddizioni che un giorno racconteremo come una delle ferite più dolorose della sua storia. È quindi giusto il coinvolgimento turco e vanno bene tutte le misure che allentano i vincoli di bilancio grazie per dar vita a una gestione collegiale delle frontiere, dell'accoglienza e dei rimpatri, anche per velocizzare le procedure di riconoscimento ed aumentare i controlli di sicurezza. È necessario giungere all'asilo politico europeo, riscrivendo così il Regolamento di Dublino e salvando l'Accordo di Schengen. Inoltre, siamo tutti molto preoccupati

Ringrazio il Presidente del Consiglio per le parole e gli impegni che ha speso sul Brennero nel suo ultimo intervento in quest'Assemblea. Siamo soprattutto preoccupati perché oggi il *land* Tirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto un rapporto di forte collaborazione, anche istituzionale, di cooperazione territoriale (GECT) dell'Euregio Trentino-Alto Adige-Tirolo, che, proprio in questi mesi a presidenza trentina, ha lanciato oltre 50 progetti di effettiva collaborazione transfrontaliera. È un laboratorio importante, che, proprio negli anni del centenario della Grande guerra, costruisce ponti e *tunnel* per unire territori prima divisi dalla guerra e che il Presidente del Consiglio stesso ha indicato come un modello per la soluzione della crisi ucraina. Anche per questo i tre Presidenti del Trentino, dell'Alto Adige e del Tirolo nelle scorse settimane hanno dato vita a un'iniziativa congiunta sia con le autorità austriache che nell'incontro con il ministro Alfano, proprio perché consapevoli che un'eventuale emergenza profughi sarebbe un problema di tutti, a prescindere dalle frontiere. È un'iniziativa che va sostenuta e merita un'attenzione particolare, proprio perché va nella direzione di una gestione collegiale, non solo da parte dei Governi, ma anche delle istituzioni locali che vengono interessate dal problema. La chiusura della frontiera del Brennero costituirebbe una grave battuta d'arresto. Per questo chiediamo tutto l'impegno del Governo italiano con le autorità austriache e in sede europea affinché questa eventualità, che oggi appare purtroppo concreta e vicina, venga scongiurata. inoltre al Governo di tenere coinvolti anche i nostri territori che hanno ribadito totale disponibilità a collaborare attivamente. Per questo sosteniamo il Governo nell'azione che sta portando avanti, con determinazione, in Europa, consapevolezza anche del fatto che davanti alla minaccia terroristica, soprattutto quando questa riesce a fare proseliti anche nel disagio che si annida nelle nostre comunità, occorre mettere in campo forti strumenti di carattere culturale e sociale, per riaffermare la centralità dei nostri valori, per combattere il malessere sociale, per garantire condizioni di vita migliori e una prospettiva diversa di futuro. È quindi giusto ricordare all'Europa che non può essere solo il luogo delle camicie di forza della burocrazia che stritolano la nostra agricoltura, la montagna, le nostre piccole e medie medie imprese; che non può essere solo il luogo di quell'austerità che ha prodotto un pericoloso smottamento del ceto medio, che ha visto la nascita di nuove forme di povertà che credevamo non dovessero più appartenere ai nostri Paesi. Credo che la linea politica che il Governo ha intrapreso nel confronto con l'Europa sia quella giusta. Il problema vero, non del Governo ma delle istituzioni dell'Unione, è che sempre più spesso sembra di essere nel gioco dell'oca, per cui anche dopo la condivisione degli obiettivi durante i vertici, all'indomani il tutto si trasforma in un gioco di distinguo, di ritardi e di mancanze, per ritornare, tragicamente, al punto di partenza, come lo stesso Presidente del Consiglio ha realisticamente ammesso. È evidente allora che l'azione deve essere intensificata e non lasciata solo sulle spalle del Governo italiano, ma deve vedere un coinvolgimento più largo di tutte quelle forze che possono aiutare l'Europa a ritrovare la strada giusta,

sono in realtà abbondantemente contenute nel mio intervento in sede di discussione, né potevamo, ovviamente, accettare la proposta di riformulazione del Governo che avrebbe, a nostro avviso, snaturato i contenuti della risoluzione Vorrei però approfittare di pochi minuti per fare una considerazione politica, anche alla luce del dibattito che ho ascoltato e delle cose che ha detto il Presidente del Consiglio, che peraltro aveva in qualche modo anticipato nel suo intervento il presidente Casini, a proposito dei rischi che vive il continente europeo in questa fase e naturalmente del clima di grande difficoltà politica e sociale e anche di paura che attraversa il nostro continente e del rischio che tale clima possa generare in Europa una serie di fenomeni nel migliore dei casi populisti, nel peggiore addirittura ispirati da movimenti di estrema destra che potrebbero rendere il quadro politico futuro molto più complesso di quello già molto difficile con il quale ci misuriamo oggi. Il punto, però, è che nell'intervento del Presidente del Consiglio - e devo dire anche in quello del presidente Casini - c'è un non detto sul quale credo bisognerebbe ragionare ed è esattamente il perché è accaduto tutto questo in tutti questi anni. È troppo comodo dire che oggi l'Europa vive questo momento di difficoltà senza però interrogarsi

abbiano cercato di gestire la crisi e di come lo abbiano fatto, evidentemente, nel modo più sbagliato possibile. C'è una totale rimozione politica degli errori clamorosi che hanno portato oggi il continente a questo tipo di situazione.

abbiamo purtroppo assistito alla completa impossibilità di mettere in campo un ragionamento su questo. troppo facili le lacrime di coccodrillo oggi. La crisi odierna dell'Europa nasce da una enorme responsabilità politica. Purtroppo questa responsabilità politica è innanzitutto delle

Signor Presidente, innanzitutto rilevo che il presidente del Consiglio Renzi ha ritenuto opportuno andare via e non partecipare alla conclusione della discussione. Rilevo anche che anche che non ha detto a quest'Aula, non ha raccontato ai senatori, pur attenti a quello che si andrà a discutere domani in Consiglio europeo, che cosa lui andrà a dire, che cosa ha realmente recepito e di che cosa si occuperà nel merito. Non parlerò della questione dell'immigrazione perché la senatrice Fattori ha esposto in modo egregio l'intendimento del Movimento 5 Stelle.

della sua azione di Governo; egli ci ha parlato di come l'economia italiana si sia riattivata a seguito dell'azione di questo Governo, di come si siano riattivati i consumi, l'occupazione e l'economia in generale; di come l'economia stia attraversando un momento di forma smagliante grazie all'azione del Governo e di queste pseudoriforme chiamate con termini inglesi per non farle capire agli italiani. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio si scontrano, però, con la dura realtà e sono proprio i fatti e i numeri di cui ha parlato anche la senatrice Lezzi - che noi citiamo nelle premesse delle nostra risoluzione che danno forma e sostanza al fallimento di questo Governo e alla mistificazione circa la situazione del nostro Paese in Europa, che di certo non ha terreno fertile. Il dato è che l'Italia è sull'orlo di una bocciatura. La riunione dell'Eurogruppo dello scorso 7 marzo è solo l'ultimo degli ammonimenti e delle preoccupazioni che gli attori comunitari rivolgono al nostro Paese. Il Governo di fatto non sta rispettando le regole europee in ambito di risanamento del debito e non basterà, quindi, la tanto vantata flessibilità ottenuta in sede di contrattazione europea per evitare il rischio di un giudizio negativo. È facile spiegare questa bocciatura. Se le risorse finanziarie accordate al nostro Paese fossero veramente state utilizzate per far ripartire la nostra economia, non staremmo qui a discutere dell'ennesima bacchettata sulle mani dell'Italia da parte dell'Unione europea. Da mesi il Governo si fa bello; si parla dell'incremento del PIL: prima lo 0,9 per cento in più, poi lo 0,7;

Ciò che ha spinto questa miseria crescita, vantata dal Governo, in realtà non è il *jobs act*, ma sono fattori congiunturali, vale a dire eventi esterni alla nostra economia: il calo del prezzo del petrolio, la svalutazione dell'euro e il *quantitative easing*; e questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma è agli occhi di tutta l'Europa. Inoltre, il calo dei costi di produzione dei beni di consumo causato del calo del costo dei fattori produttivi senza un adeguato sostegno al reddito e al rilancio dei consumi fa sì che oggi in una condizione economica problematica: quella della deflazione. Questo lo confermano gli ultimi dati ISTAT di oggi, e non di un anno fa. Ancora, il presidente Renzi sostiene, che l'incremento occupazionale in effetti c'è stato. mettersi d'accordo con se stesso: un mese fa in quest'Aula parlava di 756.000 contratti di lavoro a tempo indeterminato. parla di 950.000 contratti. Poi dice che sono trasformazioni; poi parla di precari che hanno ricevuto la possibilità di avere un contratto di lavoro trasformato a tempo indeterminato. In verità, la maggior parte delle trasformazioni a volte è stata frutto di frodi, e questo è stato ampiamente discusso anche in Commissione lavoro, anche attraverso la mia interrogazione e con le risposte del Governo che ha ribadito che non riesce a controllare le frodi. sono un incremento occupazionale bassissimo a fronte di 12 miliardi spesi. 20 miliardi strutturali spesi che non hanno avuto alcun incentivo sui consumi italiani. Qui parliamo di almeno 32 miliardi sperperati anziché fare investimenti strutturali, investimenti sulle

potere contrattuale in Europa e non può chiedere flessibilità, perché a fronte della richiesta di flessibilità non corrispondono vere riforme che hanno prodotto una reale crescita del nostro Paese.

facciamo i migliori auguri al presidente Renzi, in vista del Consiglio europeo di domani, sebbene sia certo che affronterà per l'ennesima volta questioni che l'Europa non riesce a risolvere. Non ho alcun dubbio: la sfida che giocherà su immigrazione, occupazione e crisi economica sarà solo un'altra missione impossibile. Il delicato momento, caratterizzato da massimi flussi, rende difficile coniugare il principio della libera circolazione con quello della sicurezza e del controllo dei migranti. Obiettivo dell'Unione europea in questo momento è quello di salvare l'accordo di Schengen, ma le tematiche migratorie debbono essere reinserite in un quadro europeo coeso e logico e non, ahimè, in uno scacchiere internazionale frammentato, in cui sei Paesi europei hanno sospeso Schengen: Austria, Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia e Germania. La gestione dell'immigrazione è un tema scottante, pervade le politiche di ogni Stato dell'Unione e porterà a lievitare i costi già esosi. Ricordo, infatti, che la stima degli oneri ulteriori per la chiusura delle frontiere interne Schengen, laddove si dovesse verificare, ammonta a 1.400 miliardi di euro in un decennio, per cui questa sciagura veramente non ce la possiamo permettere. Emblematico, in tal senso, il voto di domenica in Germania che ha evidenziato, premiando i partiti euroscettici, le preoccupazioni della gente comune verso un'accoglienza senza regole. Al contrario, il perseguimento della Europa economica e monetaria ha necessità di abbattere le frontiere per le persone e le merci. È necessario, pertanto, tracciare un quadro europeo logico, che prenda le distanze da una politica ondivaga rispetto a un tema che, già un anno fa, segnava l'evidenza di tutta la propria problematicità. Ricordo, a tal proposito, come ha detto poc'anzi il presidente Renzi, che in poco meno di un anno l'azione della Unione europea in materia di immigrazione ha visto ben quarantuno incontri e riunioni ai massimi livelli in Europa e ben sedici provvedimenti differenti adottati.

Questo ha fatto in modo che dal fenomeno delle migrazioni, dalla Siria e da altri paesi dell'Est, fossero coinvolti anche i Paesi della Mitteleuropa e del Nord del vecchio continente. Così come hanno indotto tutti i Paesi balcanici a chiudere materialmente le proprie frontiere. Ritengo che l'appello del presidente Renzi a non costruire nuovi muri difficilmente potrà essere accolto da tutti i Paesi europei, giustamente allarmati da questa immigrazione incontrollata. Speriamo che con la sua dialettica, così come ha cercato di convincere oggi noi che tutto andasse bene in Italia, riesca a ottenere questa

la politica non può essere ondivaga: prima dura, poi morbida e accogliente, facendo varcare i propri confini ad oltre un milione di profughi, e poi mostrando il pugno di ferro e, oggi, di fatto, bloccando le frontiere con la Turchia, non in maniera ma invitando la Turchia a mantenere, con 564 milioni di euro di investimenti, i profughi all'interno del territorio turco. Naturalmente la Turchia questo lo sa, prende 564 milioni dalla Germania, dalla Germania, 280 milioni dall'Italia e adesso, siccome i soldi non gli bastano più, probabilmente chiederà il raddoppio: pagheremo tre miliardi di euro il trattenimento dei profughi siriani e di altri Paesi all'interno della Turchia. Mi auguro comunque che il Consiglio europeo di domani, occupandosi dei temi della migrazione, non trascuri i temi dell'occupazione, della crescita e della competitività,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo ha presentato e naturalmente voterà la risoluzione con la quale vengono approvate le comunicazioni svolte oggi in questa sede dal Presidente del Consiglio. Ma nel rispetto di quello che dovrebbe essere lo spirito autentico di queste occasioni, troppo spesso fuorviato da elementi di polemica politica, io vorrei tornare su alcune questioni che sono state enunciate dal Presidente del Consiglio e che costituiscono, costituiscono, mi pare, il cuore di quelle che saranno le sedute del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo. Vorrei cominciare, raccogliendo anche il senso di un dibattito che si è svolto qui nel pomeriggio con alcuni interventi che ho particolarmente apprezzato (mi riferisco all'intervento del presidente Casini), da un'affermazione di quest'ultimo circa la necessità di superare la crisi europea provocata

non soltanto se stessa e la propria politica, ma lo spirito e l'anima dell'Europa, non riconoscibile oggi da chi guardasse la quantità di recinti, fili spinati e muri che dividono gli Stati europei, uniti nell'Unione europea, e a chi guardasse i campi profughi al confine con la Macedonia. Se arrivasse un alieno certamente stenterebbe a riconoscere in quello che vede quello che fu il sogno dei Padri fondatori dell'Unione. Voglio venire al punto forse più difficile e spinoso della questione, che è quello che riguarda l'accordo con la Turchia e la soluzione che così si dà al flusso migratorio che proviene da quella parte del mondo, non alla questione migratoria. Sono due questioni L'una, quella del flusso migratorio, è contingente e frutto anche degli errori dell'Europa; l'altra è certamente di più ampio respiro e di una qualità che ancora, neanche con l'Agenda europea e con la sua applicazione, siamo riusciti in nessun modo ad attingere. Partiamo da un'affermazione semplice: oggi dobbiamo fare l'accordo con l'Europa perché si sono chiuse le rotte balcaniche e le frontiere dei Paesi europei, perché l'Europa non è più l'Europa di Schengen, altrimenti non avremmo il bisogno di ricorrere alla Turchia, peraltro con qualche rischio come l'intervento del senatore Mauro, che ho apprezzato, ha messo Ma come fare a riaffermare nell'accordo necessitato con la Turchia, che il Presidente del Consiglio dice che non faremo a tutti i costi, quello spirito e senso dell'Unione europea di cui parlava il presidente Casini? Ora, se noi guardassimo la cosa da fuori, potremmo dire che il trasferimento in Turchia dei migranti regolari che si trovano sulle isole greche o che stanno transitando sulla rotta per la Grecia potrebbe astrattamente integrare un'ipotesi di respingimento, e sappiamo che il divieto di respingimento è ormai *ius cogens* rispetto al diritto internazionale consuetudinario. Ma, come sappiamo, la questione può essere superata da quanto è previsto nel regime comune in materia di asilo In questa disciplina si distinguono i Paesi terzi sicuri, i Paesi terzi europei sicuri e i Paesi di origine sicuri. La Turchia non è ancora un Paese terzo sicuro; in realtà, non è neanche un Paese di origine sicuro. Questo significa che ciò che dobbiamo chiedere al tavolo del Consiglio europeo è che nell'accordo si faccia esplicito riferimento all'articolo 38 della Direttiva Direttiva Procedure, e si chieda alla Turchia di osservare esattamente quelle condizioni che si prevedono e che devono essere soddisfatte perché un Paese venga considerato sicuro. Questo a prescindere dal fatto che la Turchia partecipi all'Unione europea e a prescindere dal fatto che la Turchia abbia firmato la Convenzione di Ginevra perché, come sappiamo, la applica soltanto per i richiedenti asilo che provengono dai Paesi europei. Questa richiesta che io traduco, dall'intervento del Presidente del Consiglio, nel senso che non faremo l'accordo a tutti i costi e non permetteremo che questo accordo cancelli e calpesti i valori e i principi dell'Europa,

Sappiamo, peraltro, che l'accordo prevede un reciproco obbligo di reinsediamento (e qui cito anche il risultato del lavoro della 1a Commissione). Le operazioni di reinsediamento e di ricollocazione non sono andate non sono andate a buon fine e hanno avuto risultati assolutamente ridotti rispetto agli impegni che l'Agenda europea aveva assunto (addirittura rispetto a quelli che, più precisamente, aveva assunto con riguardo alla Grecia e all'Italia) per una ragione fondamentale. che la ricollocazione e il reinsediamento non hanno funzionato e non possono funzionare tra Turchia e altri Paesi europei se non si affronta l'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio europeo del 17 e del 18 marzo, cioè la revisione dell'accordo infatti fin troppo semplice dedurre che i soggetti richiedenti asilo non hanno nessuno voglia di essere ricollocati o reinsediati in altro luogo diverso da quello nel quale aspirano a vivere, probabilmente all'interno di una comunità della stessa provenienza e all'interno delle loro stesse famiglie già espatriate. Le ultime due questioni sulle quali voglio tornare, secondo me non possono più essere escluse dal tavolo della discussione del Consiglio europeo. La prima è quella che riguarda un piano di integrazione europea per quanto riguarda i minori non accompagnati: circa 70.000 nel 2015, con grande affluenza nelle Regioni del Mezzogiorno. C'è un dato tragico. Si tratta Si tratta di giovani maschi, prevalentemente, tra i quindici e i diciassette anni. Oltre la metà di loro, dopo l'identificazione, risulta irreperibile. Non è ammissibile che l'Europa si disinteressi del destino di questi ragazzi.

studiare la questione africana e organizzare un *summit* europeo che si riunisca in più sessioni per lo studio, non soltanto dei flussi migratori provenienti da quei Paesi, ma delle condizioni di quei Paesi, degli interessi economici europei in quei Paesi,

nella mia Commissione con il lavoro dei colleghi e con la partecipazione di tanti esperti). Prendiamo soltanto ad esempio due Paesi: da una parte la Germania e dall'altra parte la Nigeria. Due grandi Paesi, un Paese europeo e un Paese africano. Nel 2050, la popolazione della Germania diminuirà dal 16 al 17 per cento: sono decine di milioni di persone. La popolazione della Nigeria crescerà del 121 per cento. Ma voi davvero credete che li possiamo fermare Come vedete, troppo alta deve essere l'ambizione europea e del mondo nella gestione di questo fenomeno e noi abbiamo fortemente apprezzato lo spirito con il quale il Presidente del Consiglio qui ha aperto la sua relazione e il modo con cui in questi mesi ha continuato non soltanto a sostenere la posizione dell'Italia, ma anche la posizione di un'Europa consapevole, lucida e forte nell'affrontare un problema che non è il cambiamento dei tempi. Non stanno cambiando i tempi, sta cambiando un'epoca. in linea con la prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

*(M5S)*. Signora Presidente, probabilmente c'è stato un disguido. Chiediamo la votazione per intero e non per parti separate.

Signora Presidente, colleghi senatori e senatrici, l'educazione alla legalità costituisce un valore irrinunciabile per la formazione di cittadini consapevoli in una società rispettosa dei diritti fondamentali È dunque indispensabile costruire un percorso di condivisione della memoria tra gli italiani, in particolar modo tra i giovani, sulla storia recente della Nazione, caratterizzata da enormi sforzi e sacrifici anche estremi volti ad affrancare l'Italia dalla presenza di tutte le mafie. La lotta a tutte le mafie è elemento essenziale per la costruzione di una nuova Italia e le istituzioni scolastiche rappresentano strumenti strategici e fondamentali per radicare questa memoria fra le giovani generazioni, come base su cui costruire un percorso di consapevolezza e radicare i valori di giustizia e legalità, in difesa delle istituzioni democratiche. Il disegno di legge in esame propone di istituire la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è il simbolo della speranza che si rinnova. Dal 1995 ogni 21 marzo si celebra la Giornata della memoria e dell'impegno: memoria per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie e impegno perché il miglior modo per fare memoria e per respingere le retoriche della memoria è quello di impegnarci ancora di più. circa 900 i nomi di vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle Forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali sono morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. A questa data l'associazione antimafia Libera ha già da anni attribuito valenza simbolica, impegnandosi in attività volte a mantenere vivo il ricordo delle vittime innocenti della mafia. Il prossimo 21 marzo si svolgerà a Messina e, in contemporanea, in tanti luoghi in tutta Italia la XXI Giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie intitolata: «Ponti di memoria, Luoghi di impegno». Quella memoria, come sottolineato dal fondatore di Libera don Luigi Ciotti, «che diventa responsabile e che dal ricordo del passato può generare impegno e giustizia nel presente». La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, nello stesso giorno e alla stessa ora, unirà Messina con i tanti luoghi in tutta Italia e non solo. Quest'anno, infatti, la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia cambia connotazione e si allarga anche verso alcune capitali europee come Berlino, Losanna, Zurigo e Bruxelles, dove sono previste numerose iniziative in concomitanza con quelle nel nostro Paese. Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli enti locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti cittadini, insieme alle centinaia di familiari delle vittime, si ritroveranno in tanti luoghi per ricordare, nome per nome, tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il Paese un ideale filo di memoria, quella memoria responsabile che, dal ricordo, può generare azione propulsiva per il futuro. L'istituzione di tale Giornata rappresenta un'occasione per restituire centralità al tema della lotta alle mafie, per promuovere la cultura della giustizia e della legalità, per responsabilizzare i giovani e stimolarli a un impegno personale nella difesa dei valori della convivenza civile. In particolare, durante tale Giornata potranno essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e iniziative volte a costruire una memoria delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e repressione Ai giovani deve essere testimoniato costantemente l'esempio di Falcone e Borsellino, così come deve esse ravvivata la fiamma della grandezza morale e del sacrificio estremo di don Giuseppe Diana. Queste figure non devono divenire con il tempo semplici nomi e il loro agire quotidiano e la loro levatura morale non devono essere dispersi con lo scorrere del tempo, che porta ogni cosa nell'oblio. Perciò ben vengano manifestazioni e cerimonie che permettano ogni anno di rinvigorire la convinzione che nulla è stato vano, nemmeno il sacrificio di una vita umana. Dal punto di vista politico-istituzionale, molto è stato fatto in questa legislatura per contrastare ogni forma di fenomeno mafioso. A maggio 2015 il Parlamento ha approvato l'inserimento nel codice penale degli ecoreati. Devastazione dei territori, inquinamento, interramento e scarichi di rifiuti tossici diventano per la prima volta in Italia reati punibili per legge e non colpe vaghe, che troppo spesso hanno visto impunite aziende e mafie responsabili dell'avvelenamento delle nostre terre. Si è giunti ad una vittoria parziale, ma importante, a fronte di una battaglia ventennale contro le ecomafie e per la riconversione ecologica dell'attuale modello di sviluppo; una battaglia che non si arresta e che continua invece a radicarsi nei territori e a rivendicare avanzamenti. Nella prospettiva della ripresa economica del Paese e del Mezzogiorno in particolare, bisogna continuare nell'azione di contrasto alla mafia quale attore economico. La criminalità organizzata è, infatti, un attore economico non di poco rilievo, come dimostrano i dati relativi ai ricavi delle mafie, che equivalgono ad alcuni punti di PIL, con 25 miliardi di euro di ricavo dal solo traffico di stupefacenti, fino alle confische per 1,3 miliardi in un solo anno. un attore che compromette la ripresa, con un effetto freno soprattutto sul Mezzogiorno, rilevato anche dalla Banca d'Italia. Sono mafie che mutano, che sono in continua evoluzione. Le più recenti evidenze investigative dimostrano la loro capacità di insinuarsi nel tessuto economico, politico e istituzionale, poiché il metodo mafioso non è più affidato al solo uso della violenza, ma anche all'utilizzo sistematico dell'arma della corruttela. In questa legislatura, è stato introdotto l'importante reato di autoriciclaggio e rivisto quello di scambio elettorale. È ora necessario rafforzare la politica e la legislazione di contrasto non repressivo, intervenendo su alcune gravi criticità che ancora si registrano nella gestione e nella destinazione dei beni e delle aziende sequestrate alle mafie. Ridarli alla società e ai territori, facendone leva di sviluppo, è un'occasione di riaffermazione positiva della legalità, oltre che di fondamentale rilancio economico e sociale. Sprecare questa occasione è un *boomerang* per lo Stato. Per questo, nel piano nazionale delle riforme contenuto nel DEF del 2015, è stata inserita la definizione di una strategia nazionale di valorizzazione dei beni confiscati. Occorre migliorare la disciplina legislativa e coordinare gli sforzi di tutte le amministrazioni centrali e territoriali impegnate su questo fronte, in sinergia con associazioni come Libera. ora stiamo aggiungendo un altro tassello. L'istituzione della Giornata per il ricordo delle vittime di mafia spero sia l'occasione e anche il pretesto per mettere in pratica le parole di Peppino Impastato che, dinanzi alla rassegnazione della sua gente, diceva: «Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. (...) È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore». Questa Giornata del ricordo dovrà infondere tutto questo nei giovani: attraverso la conoscenza del passato, avere la tenacia di non rassegnarsi e continuare a immaginare con curiosità e stupore un mondo migliore.

E, quindi, il voto è abbastanza scontato. Devo dire che c'è stata una grande partecipazione, anche in Commissione, durante la discussione di questo disegno di legge e un contributo decisivo è stato dato non soltanto dal Gruppo del PD, attraverso

qui in Aula dai colleghi del PD. Esse saranno soprattutto rese esplicite durante la dichiarazione di voto, alla quale noi annettiamo particolare importanza, come per tutti i provvedimenti.

- si sono prese un po' le distanze dal tema. In alcuni interventi si è parlato di altro, cosa assolutamente legittima, ma in questo momento mi sembra opportuno cogliere l'occasione per riportare la nostra riflessione sul tema in maniera specifica. Intanto c'è un dato da rilevare: siamo alla vigilia del 21 marzo e

ha bisogno di un riscatto e di una partecipazione collettiva, nella quale si sappia rinunciare al contributo di sangue degli eroi. Nasce così Libera, per evitare che si debbano avere questi momenti solenni, spesso fondati sul sangue

ruolo svolto negli anni, sa bene quanto quelle morti abbiano cambiato la coscienza civile di quella Regione. Lo ricordava anche un procuratore della Repubblica, qualche giorno fa,

per ricordare e dare un messaggio di responsabilizzazione della società e delle istituzioni, che devono lavorare per creare consapevolezza e coscienza civile, evitando che ci siano morti ulteriori. Esse nascono, però, anche con uno spirito molto particolare, che dobbiamo rinnovare. Perché si leggono gli elenchi

ho partecipato alla prima manifestazione di Libera, scrivendo in quell'elenco i nomi di quattro morti che, per la mia città, hanno segnato il riscatto. Due erano operai, netturbini, che abbiamo scritto come vittime innocenti, anche perché

di cui la società può scrivere che sono vittime di mafia e, quindi, ovviamente vittime senza macchia. È vero che bisogna avere pietà per tutti i morti, ma la storia dell'antimafia si deve cementare e costruire sulla storia degli innocenti e delle vittime che continuano a esserci.

tutti i nomi di persone che hanno travolto intere famiglie sul territorio, che hanno educato e potranno continuare a educare i nostri giovani a una cosa molto semplice: la mafia porta soltanto morte,

per evitare di continuare a chiedere ai nostri magistrati, ai nostri poliziotti, alle persone perbene di vivere con la paura della mafia. Noi dobbiamo invece custodire questi valori e garantire a

di dare il nostro piccolo o grande contributo - che dir si voglia - al contrasto della criminalità organizzata e al radicamento dei valori della legalità e dell'antimafia.